Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici Il presidente della 9a Commissione permanente, senatore De Carlo, riferisce sui lavori delle Commissioni riunite 8a e 9a circa 550 emendamenti e subemendamenti. Siamo ad un ottimo punto. Siamo in attesa solamente di ricevere pochissimi pareri da parte del MEF su emendamenti che, grazie anche al lavoro di grande raccordo del

sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche, finanziarie e investimenti strategici

certamente irrituale che inizi la discussione generale in assenza del testo di cui si parla in Aula: questo è il primo elemento. Ancor più irrituale è che si chieda ai Gruppi di presentare gli emendamenti sulla base di una bozza del testo A, che poi potrà cambiare a seconda delle risultanze della Commissione bilancio che nel frattempo si è espressa. Chiedo quindi innanzitutto che i termini per la presentazione degli emendamenti in Aula siano di un'ora a partire dalle disponibilità del testo A definitivo, ma che anche la discussione generale inizi dopo che il testo A sarà definitivo, cosa che al momento non è. La discussione generale inizierà quando il testo è pronto.

Vorrei ringraziare il collega Bergesio, per il lavoro che mi ha aiutato a svolgere come correlatore, i Presidenti delle Commissioni 8a e 9a e tutti i colleghi, anche dell'opposizione, perché il Parlamento ha lavorato come dovrebbe, esaminando 550 emendamenti, uno per uno, senza scartarne nessuno. Ovviamente questo ha portato a un prolungamento dei tempi, però devo dire che come relatori siamo estremamente soddisfatti del lavoro compiuto, perché questo provvedimento, che è arrivato già corposo dal Governo, è stato enormemente arricchito dall'intervento delle Commissioni riunite 8a e 9a. Ringrazio pertanto tutti i colleghi per il buon lavoro che è stato svolto.

In Commissione ho avuto modo anche di sentire nei loro interventi i rappresentanti delle opposizioni cercare di sminuire la portata di questo decreto-legge. Qualcuno ha sostenuto addirittura che il testo conterrebbe troppi argomenti, io onestamente sarei preoccupato del contrario: sarei preoccupato se ne contenesse pochi, perché purtroppo non sono pochi i problemi che sono stati lasciati in eredità a questo Governo. A differenza del passato, in cui si fuggiva davanti ai problemi, questa maggioranza invece affronta con determinazione le criticità che affliggono la Nazione. Ho ascoltato in Commissione anche il solito argomento, ossia che è passato un anno dalle elezioni. Certamente è passato un anno in cui tutti si sono resi conto che c'è stato un netto cambio di passo rispetto al passato anche i più scettici si sono dovuti ricredere, constatando che con il presidente Meloni c'è un Governo politico che si assume la responsabilità delle scelte. abbiamo fatto scelte molto importanti. Ci siamo occupati del caro energia, che rischiava di mettere in ginocchio imprese e famiglie ed è un argomento sul quale il Consiglio dei ministri qualche giorno fa è tornato stanziando ulteriori 1,3 miliardi di euro per attenuare gli effetti del rialzo dei prezzi energetici sulle fasce più deboli. Ci siamo occupati del reddito di cittadinanza e di sanare le criticità del PNRR. Abbiamo affrontato il tema del superbonus, una legge scritta male e applicata peggio, che ha reso possibili truffe e messo in difficoltà le imprese e i conti dello Stato, con un buco di 140 miliardi. Anche oggi in Commissione i rappresentanti delle opposizioni sono tornati su questo argomento e io consiglio loro vivamente di smetterla di fare gli esperti su questo tema, perché, quando hanno avuto responsabilità e modo di occuparsene, hanno fatto un pasticcio di portata epocale. Potrei continuare per ore, parlando anche dell'autorevolezza riacquisita dall'Italia grazie al presidente Meloni a livello internazionale, ma mi fermo qui. Non sfidateci però sui risultati di questo primo anno, perché non abbiamo paura del confronto, che ci vede vincenti. *asset* è in linea con l'impegno di questo primo anno, contiene molti argomenti e vi consiglio vivamente di leggerlo con attenzione, perché racconta la determinazione del Governo a stare vicino a cittadini, imprese ed enti locali. Con questo provvedimento ci schieriamo al fianco dei cittadini per tutelarli dalle speculazioni, contrastando il caro voli, che ha portato aumenti medi nel periodo estivo anche del 40 per cento, con punte del 70, a danno soprattutto dei collegamenti con le isole. Un provvedimento necessario anche secondo il parere dell'ENAC. Questo è un decreto che si occupa di contrastare le delocalizzazioni delle grandi imprese, portando da cinque a dieci anni il termine entro il quale le aziende che hanno ricevuto agevolazioni, se decidono di delocalizzarsi, sono tenute a restituire l'incentivo preso. Tradotto: se lo Stato italiano ti aiuta con incentivi per insediare la tua azienda sul nostro territorio, in Italia ci rimani almeno per dieci anni. decreto che si occupa di aiutare le imprese agricole che hanno subito danni da peronospora alle produzioni viticole, inizialmente con un fondo di un milione di euro, che in Commissione abbiamo portato a 7 milioni. Anche qui, una risposta tempestiva tempestiva e importante del ministro Lollobrigida *(Applausi)*, e desidero ringraziare il presidente De Carlo, primo firmatario di questo emendamento. È un decreto che aiuta i Comuni in stato di dissesto finanziario, con un'anticipazione di liquidità fino a un importo massimo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. È un decreto che racconta l'impegno del Governo ad aiutare i piccoli Comuni per gli interventi di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti di loro competenza. Ditelo ai vostri sindaci che siete in disaccordo con questo provvedimento. Nel decreto *asset* troviamo anche il coraggio di introdurre la tassa sugli extraprofitti delle banche, derivanti non da investimenti fatti dagli istituti di credito, ma dall'aumento dei tassi di interesse avviato dalla Banca centrale europea per combattere l'inflazione. Il testo iniziale è stato migliorato e ora le banche possono scegliere se pagare il 40 per cento dei maggiori profitti o destinare l'intero ammontare degli extraprofitti a una riserva di bilancio da destinare alla concessione di più mutui alle famiglie e Rispetto al passato, in cui si usavano i soldi dei cittadini per aiutare le banche a risanare i bilanci, oggi si usano i soldi degli extraprofitti per aiutare cittadini, imprese e tessuto economico.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, anche oggi siamo chiamati a votare, secondo una modalità scorretta e dannosa per l'onore di questo Parlamento e per la democrazia del nostro Paese, la conversione in legge dell'ennesimo confusionario decreto governativo in stile azzeccagarbugli. Ormai ci troviamo regolarmente seduti tra questi banchi a votare provvedimenti raffazzonati, che rastrellano senza logica brandelli di tematiche che non hanno né capo, né coda, ma che vanno a incidere pericolosamente sulla crescita e sullo sviluppo sostenibile di questo Paese, impattando negativamente sulla vita di cittadine e cittadini. È imbarazzante che la maggioranza non abbia ancora definito un approccio strutturale per affrontare i veri problemi dell'Italia, impedendoci di entrare veramente nel merito delle questioni che la affliggono. A un anno dall'inizio della legislatura ci si limita a far passare con superficialità provvedimenti ed emendamenti bandierina, a diretto uso e consumo della maggioranza, bisognosa di strumenti per giustificare la sua inconsistente politica, in difficoltà rispetto alle vere sfide e alle priorità cui siamo cui siamo chiamati a rispondere. Da un anno a questa parte, il *modus operandi* della maggioranza del centrodestra non è più una semplice coincidenza, ma una pratica politica intenzionalmente opportunista e inefficace, che in nessun modo risponde alle esigenze che gli italiani ci chiedono urgentemente di affrontare. *asset*, che oggi stiamo fingendo di esaminare, le cui sorti erano già ben chiare dalle prime discussioni farsa cui abbiamo assistito in Commissione, confluiscono una miriade indistinta di disposizioni coriandolo, che, spaziando dal settore dei trasporti a quello della pesca ed arrivando persino a eliminare i tetti degli stipendi dei dipendenti facenti parte della società partecipata dello Stretto di Messina, risultano infarcite senza pudore di emendamenti che nulla c'entrano con gli articoli proposti. Questo calderone informe di norme ci impedisce, anche solo da un punto di vista logico tematico, di condurre un'analisi seria e concreta degli interventi proposti, penalizzando, di fatto, il mondo fuori, l'Italia, che si trova a subire l'ennesimo pasticcio politico. Qui, un grande assente, però, c'è. Anche questa volta, il Governo non ha messo in cima alla propria agenda le politiche di contrasto ai danni causati dal cambiamento climatico. Anche per questo provvedimento legislativo la dimensione della sostenibilità ambientale è un elemento inesistente. Sul famoso superbonus del 110 per cento, su cui si sta conducendo una irresponsabile campagna denigratoria ai danni di imprese e cittadini, non si è pensato di apportare interventi migliorativi su quanto effettivamente è risultato non aver funzionato nella sua applicazione. Si è, invece, deciso di peggiorare

il Governo è infatti intervenuto con una sciabolata, contribuendo ad aggravare la crisi che ha già investito l'intero settore edile ed una parte della società, con il dramma dei cantieri fermi e quello delle famiglie che hanno avviato lavori condominiali. Il Governo aveva poi ben pensato di tassare gli extrautili delle banche, a detta del ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Salvini per aiutare famiglie e imprese colpite dall'aumento dei tassi; salvo poi stravolgere completamente la disposizione e ingranare subito la retromarcia. A questo punto, la maggioranza ha pensato bene di avventurarsi sul tema della caccia, che con questo decreto *asset* non c'entra assolutamente nulla e, soprattutto, non ci pare rientri nelle urgenze del Paese, come invece la necessità di sostenere concretamente l'Emilia Romagna e le altre Regioni colpite da eventi climatici estremi; come quella di mettere in sicurezza il nostro territorio, di migliorare le condizioni di lavoro e di affrontare seriamente i problemi della sanità in Italia. Nel decreto oggi in discussione, nella parte recante misure urgenti per le produzioni viticole, che a logica comune ci si aspetterebbe essere relative al tema dei vitigni e della loro coltura, avete maldestramente inserito delle insensate modifiche per la pratica della caccia, scavalcando peraltro il divieto dell'Unione europea di utilizzare le cartucce al piombo nelle aree cosiddette umide. umide. Tanto per capirci, volete dare il via libera alle cartucce al piombo in laghi, torbiere, fiumi, stagni, lagune, valli da pesca, paludi, litorali con le acque marine e costiere, prevedendo una sanzione irrisoria in caso di violazione pensando di evitare o di aggirare il rischio di nuove procedure di infrazione comunitarie, che già sottraggono milioni di euro alle casse dello Stato, risorse economiche di cui il Paese ha estremamente bisogno. È palese che poco importa al Governo che le cartucce siano ambientalmente dannose a causa dell'inquinamento prodotto dal piombo sulla biodiversità e sulla salute delle persone. pensi solo agli stessi pallini di piombo che finiranno sulle nostre tavole. Evidentemente - ci viene da dire - il centrodestra le digerisce meglio. Ma tant'è. Per il Governo era prioritario proporre l'eliminazione del potere dei giudici amministrativi in caso di ricorsi sui piani venatori e il depotenziamento definitivo dell'ISPRA per estendere senza limiti il calendario venatorio. Il tempestivo intervento delle associazioni ambientaliste che hanno pubblicato un comunicato stampa congiunto, indirizzato al presidente del Senato La Russa, per denunciare il fatto e l'improponibilità di questi emendamenti, ha costretto la maggioranza a fare un irrisorio passo indietro. Riteniamo preoccupante che si debba delegare anche alla società civile il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento del Senato e sul rispetto dei parametri costituzionali previsti per la conversione in legge di un decreto governativo. A questo proposito giova ricordare che l'articolo 97 del Regolamento del Senato indica come improponibili gli emendamenti estranei all'oggetto della discussione. Altrettanto improponibile riteniamo la proposta di articolo a prima firma del Presidente della 9a Commissione che ci restituisce perfettamente la fotografia del vostro modo di fare politica. Nella parte recante misure per la ricerca e lo sviluppo nella microelettronica si inserisce un'ulteriore disposizione nella quale si autorizza il taglio di alberi e boschi. L'*incipit* di tale articolo chiarisce, senza mezzi termini, l'intenzione del Governo di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera foresta-legno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane, anche potenziando la possibilità di approvvigionamento della materia prima. Serve, insomma, legno, serve tagliare alberi e boschi. Abbiamo una forte perplessità rispetto a questa norma; ne monitoreremo gli effetti applicati per essere sicuri che le semplificazioni ora introdotte non si traducano in una gestione disinvolta del patrimonio boschivo, al solo fine di sviluppare la filiera foresta-legno. Sarebbe questo uno schiaffo al nostro Paese colpito fortemente dal dissesto idrogeologico. Ieri sera mi è stato detto dalla maggioranza che questa è democrazia. Questi sono giochi di forza alle spalle degli italiani; giochi condotti, a nostro parere, senza rispetto dei parametri costituzionali previsti per la conversione in legge di un decreto governativo di urgenza e senza rispetto della corretta applicazione del Regolamento del Senato. Giochi che in una sana democrazia non devono trovare spazio.

la legge di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante disposizioni urgenti a tutela degli utenti in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici, pone alcuni interrogativi - qualora ce ne fosse ulteriore necessità, Presidente - sul rispetto della Costituzione e delle istituzioni, con particolare riferimento al ruolo del Parlamento e sulla capacità di questo Governo di intervenire nel nostro ordinamento. La disomogeneità dei decreti-legge è un sintomo di assenza dei presupposti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 e, badi bene, Presidente, non lo dice il senatore Nave, ma la Corte costituzionale. Il contenuto del decreto-legge, che definire *omnibus* è un eufemismo, è un coacervo di problematiche sorte durante l'estate che, non essendo stati in grado di affrontare in maniera sensata e con efficienza, avete inserito frettolosamente in un calderone che non ha né capo né coda. Si passa dai taxi agli extraprofitti, dove poi si è dovuto aggiustare il tiro per non incorrere in un vizio di legittimità costituzionale, passando per le produzioni vitivinicole, gli investimenti strategici, il caro voli; insomma, chi più ne ha, più ne metta. Presidente, lungi da me sminuire i problemi che questo decreto-legge aveva in mente di risolvere. Sono problematiche sentite che gravano sui cittadini, ma questo - come diciamo da tempo - non è modo di operare. Questa confusione di materie il solo effetto di creare delle problematiche di natura operativa e istruttoria all'interno delle Commissioni. Qualcuno della maggioranza mi dovrà spiegare in che maniera si pensa di eseguire un'istruttoria adeguata se la 9a Commissione, competente per attività produttive, turismo e agricoltura, viene ritenuta competente in materia di tassa sugli extraprofitti. Capisco che la vostra concezione del Parlamento è quella di una scatola vuota, come se il Parlamento dovesse solo ratificare le vostre decisioni, attribuendo a questo un mero ruolo notarile. Ma qui, Presidente, si è veramente superato ogni limite. Questi aspetti, ancorché preoccupanti, non sono l'apice del vostro scarso senso istituzionale: l'apice si è raggiunto con gli emendamenti del Governo, laddove questi venivano pubblicati una settimana dopo che ne fu data notizia alle agenzie di stampa. Ancora, qui si avalla l'idea del partito che rappresento, vale a dire che questo non è un decreto-legge: è il vostro *spot* pubblicitario per l'estate. Ovviamente, Presidente, credo sia utile rendersi conto della gravità di far uscire gli emendamenti governativi prima sui giornali e poi in Parlamento,

Queste criticità sul vostro metodo parlano da sole: sono sintomi di un *modus operandi* oltre che inutile, fortemente irrispettoso della nostra Costituzione e dei ruoli che essa riserva alle singole istituzioni, *in primis* al Parlamento. Ma al peggio non c'è mai fine. Ora, Presidente, veniamo al merito. Chiaramente, per ragioni di tempo non posso soffermarmi su tutti gli articoli, ma su due in particolare bisogna intervenire: il caro volo e il tema TIM. L'articolo 1 del decreto-legge partiva con degli errori di fondo clamorosi, motivo per cui siete intervenuti autocorreggendovi, però facciamo un passo indietro. Anzitutto dobbiamo constatare che la destra, benché in audizione al Senato i commissari di maggioranza facessero la voce grossa con le compagnie aeree, ha ceduto ai ricatti. Il ministro Urso ha fatto dietrofront. Si sono inventati una procedura di monitoraggio e di intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che non è chiara rispetto ai criteri da tenere in considerazione. Tra i criteri che l'AGCM può tenere in considerazione, vi è l'eventualità in cui vi sia un aumento del prezzo di vendita del biglietto e dei servizi accessori nell'ultima settimana antecedente il volo, superiore alla tariffa media del volo di oltre il 200 per cento. Per intenderci, se il biglietto viene acquistato nella settimana precedente al volo e la tariffa media è di 100 euro, qualora il prezzo praticato sia di 300 euro, l'AGCM deve tenerne conto, ma solo nel caso in cui l'acquisto venga effettuato, appunto, nella settimana. Di conseguenza, logica vuole che se il biglietto viene acquistato cinque giorni prima e il prezzo praticato è superiore al 200 per cento non vi sia alcun problema. Inoltre si parla di prezzo medio senza identificare quale sia il parametro temporale da tenere in considerazione. Anche in questo caso un esempio pratico aiuta a capire: poniamo il caso che venga ridotta l'offerta di voli come è già successo dopo le improvvide uscite del ministro Urso, facendo aumentare di conseguenza la tariffa media da 100 a 150 euro. In questo caso, stando alla scrittura della norma, un biglietto da 300 euro non sarebbe più un prezzo eccessivo, in quanto non supera del 200 per cento la tariffa media praticata. Insomma non gli riesce proprio di fare le cose bene. Da un lato, non si comprende il funzionamento della legge della domanda e dell'offerta e, dall'altro, si scrivono norme sotto dettatura delle compagnie aeree, senza rendersi conto dei danni che si producono ai cittadini. Questa frenesia di uscire sui giornali con i titoli eclatanti sta mandando a scatafascio un intero Paese. Unica nota quasi positiva è quella di aver inserito dei criteri di trasparenza per la rendicontazione delle sovvenzioni pubbliche alle compagnie aeree. Ovviamente, questa norma era già stata chiesta dalla collega Lupo del MoVimento 5 Stelle nella passata legislatura. Dico "quasi" positiva, perché in realtà i criteri di trasparenza sono stati annacquati rispetto alle richieste del MoVimento 5 Stelle. Altra nota dolente è rappresentata dall'articolo 13, che il Governo velatamente presenta come uno strumento da poter utilizzare per gli *asset* strategici del Paese, mentre è chiaro a tutti che si riferisce alla NetCo di TIM e quindi al futuro che questo Governo vuole assicurare alla rete nazionale delle telecomunicazioni, per noi *asset* strategico, appunto. Ci saremmo aspettati da un Governo di destra sovranista (a parole) l'impegno ad acquistare quote importanti della stessa per poterne indirizzare le politiche economica e industriale. Invece ci troviamo di fronte a un timido approccio, senza un piano industriale, che porterà a depauperare il patrimonio destinato a Cassa depositi e prestiti che si vuole usare per l'acquisto. A proposito, Presidente, questo è un fondo creato da Conte nel 2020 per acquistare solo il 20 per cento delle quote, lasciando la quota di maggioranza ad un fondo straniero (KKR, appunto). Eppure, narrate che nonostante tutto il Governo avrà pieno potere di decisione. Non capisco a quale manuale di diritto commerciale si faccia riferimento, per cui una società di minoranza possa poi dettare legge. Insomma, oggi è il caso di dire che da italiani sovranisti a sudditi di multinazionali straniere è proprio un attimo. *(Applausi)*. Presidente, onorevoli colleghi, oggi discutiamo del provvedimento noto come decreto *asset*, che contiene un articolato importante e complesso che incide sulla carne viva del tessuto sociale ed economico del nostro Paese. Si tratta di un provvedimento che si pone due obiettivi principali: da un lato cerca di dare risposte rapide a problematiche emergenziali ed urgenti in favore dei cittadini e delle attività economiche, problematiche alle quali il Governo non poteva sottrarsi e alle quali, infatti, non si è sottratto; dall'altro lato tenta di riportare un equilibrio e una giustizia sociale rispetto a fenomeni economici che si sono manifestati negli ultimi tempi. Mi soffermerò solo su alcuni aspetti, non su tutti, anche se sono meritevoli di attenzione ed approfondimento. Partirei proprio dall'articolo 1 del provvedimento, che tratta del caro voli aerei in determinati periodi da e verso le isole maggiori, che sancisce un principio fondamentale: non si possono consentire speculazioni insopportabili che colpiscono i cittadini nel loro diritto fondamentale alla mobilità. Si prevede, dunque, l'ampliamento dei poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sulla concreta verifica del funzionamento degli algoritmi sui quali poggiano pratiche di fissazione dinamica della tariffe dei voli quando ricorrono determinate condizioni. È una norma coraggiosa sulla quale l'Italia sta facendo scuola. Noi abbiamo un Governo che il problema se lo è posto e lo ha risolto, perché se da un lato è giusto garantire il diritto alla concorrenza delle imprese private, dall'altro ancor più giusto è tutelare il diritto alla mobilità a prezzi accessibili per quei passeggeri che subiscono svantaggi derivanti dall'insularità o da eventi calamitosi, quando non vi è la possibilità di muoversi in altro modo. Quando parliamo di divario sociale, dobbiamo tenere a mente che la mobilità è fondamentale anche e soprattutto per chi abita in un territorio come le nostre meravigliose isole e che deve avere le medesime possibilità di spostamento di qualsiasi altro cittadino italiano a prezzi giusti. Questa norma tenta di ristabilire un equilibrio quando questo viene intaccato da pratiche scorrette. Andando avanti nell'analisi del provvedimento, altro articolo particolarmente importante per lo sviluppo industriale italiano è quello che incentiva la filiera dei *microchip.* La pandemia Covid e la guerra in Ucraina hanno posto in evidenza con rilevante drammaticità le problematiche derivanti da un modello globale di approvvigionamento e produzione di beni. Le misure restrittive alla circolazione dei beni che possono derivare da pandemie, come abbiamo potuto sperimentare, o da embargo o da qualsiasi altra motivazione geopolitica hanno causato e possono causare inevitabilmente la paralisi endemica dei flussi commerciali. Quello della carenza di determinati beni è un problema che ha messo in evidenza una certa fragilità dell'Europa, Italia inclusa, che dipenda, per l'approvvigionamento di numerosi prodotti

La norma contenuta in questo decreto, che riconosce il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo della microelettronica, risponde quindi a un problema reale trasformandolo in una sfida per l'Italia. Con questa norma diamo avvio a una strategia volta ad implementare una maggiore autonomia interna rispetto alla produzione e approvvigionamento di semilavorati che sono ritenuti strategicamente essenziali per i nostri piani di sviluppo. Con questo provvedimento, il Governo Meloni incentiva la creazione di una rete di produzione in Italia di semiconduttori al fine di ridurre la dipendenza da altri Stati. È una norma che dà una risposta concreta ad un problema che ha tenuto sotto scacco molte nostre aziende in questi ultimi anni. sarò breve, ma non possiamo non parlare dell'articolo 26, cui ha accennato anche il collega Sigismondi, recante la norma sugli extraprofitti bancari. In un mercato del credito realmente concorrenziale i tassi attivi e passivi, cioè quelli che la banca chiede al cittadino sui prestiti e quelli che gli offre per i soldi depositati sui conti,

Con questa norma le banche verseranno allo Stato un'imposta straordinaria sull'extraprofitto generato nel 2023, determinato sulla differenza fra gli interessi attivi e quelli passivi confrontati con gli stessi dati del 2022. Tale imposta sarà destinata a un apposito fondo volto a finanziare il fondo di garanzia mutui prima casa e interventi finalizzati alla riduzione

che servirà a consolidare il loro patrimonio, troppo spesso debole rispetto a fenomeni finanziari nazionali e internazionali. In questo modo eviteremo in futuro che il ripianamento delle perdite delle banche ricada sui cittadini: una per tutte ricordo la vicenda del Monte dei Paschi di Siena. Mi avvio alla conclusione, dicendo che il decreto-legge in discussione è l'ennesima prova di un Governo politico che l'Italia non vedeva da dieci anni, che ha una visione su come devono andare le cose e ha una sua maggioranza solida.

pomposamente ribattezzato decreto *asset.* Dico subito in premessa che di strategico in questo provvedimento non c'è proprio nulla Anzi, esso si caratterizza non per quello che c'è, ma per quello che manca o meglio per quello che è stato annunciato

penso all'inflazione che erode il potere di acquisto dei ceti medi facendoli scivolare verso l'impoverimento; penso alle file e alle code dei cittadini in attesa di un taxi; penso ai prezzi alle stelle per raggiungere in aereo la Sicilia o la Sardegna durante l'estate - ai quali però si risponde con misure che strizzano l'occhio al consenso popolare penso alla norma sugli extraprofitti, al tetto massimo sul caro voli, alle nuove licenze dei taxi - e poi ci si rende conto che queste misure sono impraticabili o incompatibili con il quadro normativo italiano ed europeo e allora le si stralcia dal testo legislativo e le si annacqua di contenuto tanto da farle diventare acqua fresca. Dal punto di vista della comunicazione politica, di tutto ciò rimane il consenso effimero creato da qualche titolo altisonante sui giornali, in TV, sui *social,* ma dal punto di vista normativo non rimane niente.

Beninteso: su alcuni provvedimenti che erano stati annunciati, per come erano stati configurati, fortunatamente si è fatto un passo indietro. Parto subito entrando nel merito della misura più controversa: la norma sugli extraprofitti delle banche. Cerco di essere più semplice possibile, anche se la norma è delicata e complessa e non consente semplificazioni che portino alla banalizzazione dell'argomento. Qual è stata la strategia comunicativa del Governo? Prendere un problema serio, anzi serissimo, come il tema dell'impoverimento degli italiani causato dall'inflazione, e cercare di risolverlo nel modo più sbagliato possibile. Lo avete fatto non intervenendo sulla sterilizzazione delle accise sulla benzina, come fece il Governo Draghi *(Applausi)* proposto anche noi sotto forma di emendamento, per il quale ringrazio la collega Silvia Fregolent per il lavoro incessante, nonostante il caos dei lavori in Commissione. Si tratta di un emendamento che la maggioranza ha respinto e per il quale vi prendete la responsabilità davanti agli italiani, che oggi pagano il pieno di carburante molto di più di quanto lo pagavano un Lo avete fatto non intervenendo sulla proposta di salario minimo avanzata dalle opposizioni, per il quale ancora aspettiamo fiduciosi la vostra controproposta, ma intervenendo con gli appunti di Giorgia con data 9 agosto: «Stiamo registrando utili record. Abbiamo deciso di intervenire introducendo una tassazione del 40 per cento sulla differenza ingiusta del margine di interesse. Le risorse che arriveranno andranno a finanziare misure di sostegno a famiglie e imprese in difficoltà per l'alto costo del lavoro». Wow, modello Robin Hood: togliamo i soldi alle banche ingorde e cattive e li diamo ai poveri. Wow. Vedi ad avere una Presidenza del Consiglio forte, che finalmente attacca i poteri forti e le banche? banche? Onorevoli colleghi, mi dite cortesemente in quale disposizione di questo testo gli appunti di Giorgia sono diventati norma? Stimo la vostra intelligenza, per cui so che non mi risponderete riprendendo l'arabesca disposizione dell'articolo 26, in cui oggi le banche "possono" (non devono) scegliere se pagare un'aliquota del 40 per cento sulla differenza tra il margine che hanno realizzato, oppure se accantonare una riserva al proprio patrimonio. Dal punto di vista giuridico, bastava leggere quello che la Banca centrale europea, sulla medesima proposta che era stata avanzata dal Governo della Lituania, aveva dato, ammonendo sulla necessità di preservare la solidità patrimoniale delle banche per garantire la capacità di erogare credito. Eh sì, perché le banche devono mantenere una posizione patrimoniale adeguata per poter fungere da cinghia di trasmissione delle misure di politica monetaria all'economia in generale. Tradotto negli appunti di Giorgia: se tocchi alle banche lo 0,1 per cento del totale dell'attivo, ma poi a causa di questo le banche non danno più mutui ai piccoli risparmiatori, non stai facendo affatto una cosa che aiuta gli italiani che sono in difficoltà.

favorire la concorrenza leale tra i vettori aerei. Avevo presentato un emendamento a firma mia e del Gruppo per dire che le compagnie aeree, come Ryanair e ITA Airways, che sistematicamente, in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, non danno la compensazione pecuniaria, oltre alla riprotezione del volo, violano la carta dei diritti fondamentali del passeggero e andrebbero sanzionate per concorrenza sleale. Voi invece che fate? Annunciate la tariffa massima del 200 per cento sulla tariffa media, senza peraltro specificare qual è l'orizzonte temporale (un giorno, un mese, un anno?) e poi, quando vi rendete conto che questa farebbe scappare i vettori aerei, la ritirate. Per non parlare delle licenze del taxi: stesso film. Problema vero: le code alle Soluzione presentata da noi: una licenza aggiuntiva a chi è già titolare, in modo da aumentare la concorrenza, senza penalizzare i tassisti di oggi, ma ciò non viene accolto. Passo avanti, passo indietro, dietrofront: mi chiedo se è rimasto qualcuno di liberale in questa maggioranza o se le parole «concorrenza leale» fanno fatica ad entrare nel linguaggio politico di una certa parte di questa maggioranza. *(Applausi)*. L'unica cosa della quale vi devo dare il merito di averci ascoltato è aver esteso non solo alla Sicilia e la Sardegna, ma a tutte le Regioni interessate, il fondo a favore degli operatori del settore turistico per i danni degli incendi. Non avete fatto un favore a noi o al Gruppo, ma avete fatto una cosa giusta per territori come ad esempio il Comune di Vieste, che ha stimato un danno ambientale di 1 milione di euro per gli incendi del luglio 2023 che hanno interessato la Regione Puglia. Temo che le risorse che avete messo su quel fondo non siano sufficienti a ristorare i danni da incendio, ma almeno apprezzo la vostra buona volontà. La stessa cosa non posso dire per quanto riguarda gli emendamenti che avevamo presentato per la ricostruzione dei territori colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna, riprendendo la legittima richiesta di tanti amministratori locali e del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. Ebbene, ci avete respinto tali emendamenti senza giustificazione. Arrivo alla conclusione. Non chiamatelo decreto-legge *asset.* Sul nostro territorio italiano scoppiano ogni giorno delle crisi aziendali: solo per rimanere nel territorio dell'area metropolitana di Bologna, penso alle lavoratrici de La Perla e ai lavoratori della Magneti Marelli, a cui sabato prossimo andremo non solo a presentare la nostra solidarietà, ma anche a spiegare quali sono le responsabilità precise che non hanno consentito lo sviluppo dell'azienda e che mettono a rischio la salvaguardia della sua capacità produttiva e dei posti di lavoro. Voi dovreste essere capaci non di decantare la sovranità nazionale, ma di esercitarla e magari di esercitare la *golden power* a tutela degli investimenti: questi sì che sono strategici per l'interesse nazionale. Allora chiamiamolo "decreto dietrofront". State attenti, la strategia di comunicazione politica può durare un po' di tempo, ma non a lungo. Mentre la nave Italia continua a galleggiare senza una rotta, senza una visione, senza una strategia, gli italiani non si fanno e non si faranno prendere in giro: non sono così sprovveduti da non capire che così ci si prende gioco di loro. Quando la loro fiducia viene tradita, il consenso effimero della comunicazione politica svanisce come d'incanto se mancano le risposte concrete ai loro bisogni, alle loro paure e alle loro speranze.

Presidente, mi rivolgo a lei per dire subito che la nave Italia veleggia verso mari sicuri e porti sicuri *(Applausi)*, e anche con l'approvazione oggi di questo provvedimento il Paese farà due passi in avanti, anche grazie al confronto proficuo che c'è stato all'interno della nostra maggioranza, che ha portato a migliorare il provvedimento. Signor Presidente, mi rivolgo ancora a lei per dire: basta, è passato oramai un anno, eppure citiamo sempre e soltanto il Governo Draghi, del quale abbiamo fatto parte anche noi, ma un anno fa. Oggi festeggiamo un anno, gli italiani hanno votato e hanno fatto una scelta netta: hanno scelto nelle urne, in maniera democratica, il centrodestra e il Governo del centrodestra. *(Applausi)*. Abbiamo oggi titolo a governare e lo facciamo non con la poesia

perché si tratta di un decreto di agosto, in un periodo in cui anche la politica per qualche giorno è andata in ferie e quindi i giornali hanno certamente dato risalto a questo aspetto. Oggi, grazie anche alle nostre proposte, andiamo a migliorare il provvedimento in esame. Sin dal primo momento, d'accordo su questa imposta; abbiamo soltanto cercato di tracciare un po' quello che poteva essere il perimetro in un momento particolare, che serviva e serve oggi a sostenere e aiutare le famiglie e le imprese

è stata migliorata la norma, con una semplice riscrittura che soddisfa tutti, perché è sì cambiata, ma alla fine abbiamo mantenuto - e l'abbiamo sempre detto - invariato il gettito dell'entrata prevista a sostegno di famiglie e imprese. È importante aver posto un

patrimonializzare una banca? Significa poter aiutare ancora di più le famiglie e le imprese. Ecco perché abbiamo migliorato e siamo tutti più contenti di approvare questo provvedimento. Altro che un passo indietro: due passi in avanti. Cambiano inoltre i beneficiari delle entrate della norma, che - come dicevo - alimentare il fondo per il mutuo della prima casa, per ridurre la pressione fiscale e per alimentare il fondo da cui attinge Mediocredito Centrale per dare garanzie di sostegno alle nostre imprese. Meglio di così io ritengo che il Parlamento non potesse fare. Lo abbiamo fatto ed è oggi nostro merito confrontarci e riuscire sempre a dare risposte agli italiani.

continuo, spropositato e così veloce, ha messo in difficoltà le famiglie. Da tempo, sin dall'inizio della legislatura, io, insieme con tutta la maggioranza e il mio Gruppo parlamentare, chiedevo di fare attenzione, perché questo momento avrebbe messo in difficoltà e quindi era necessario creare un fondo per aiutare e sostenere. Lo abbiamo fatto nella manovra finanziaria dello scorso anno, quando abbiamo stabilito, attraverso lo *switch* automatico alle banche, che i clienti che avevano sottoscritto dei mutui a tasso variabile potessero, senza assolutamente alcun tipo di documentazione o pratica, switchare il mutuo da tasso variabile a tasso fisso. Abbiamo messo

Voglio ricordare l'articolo 3, che riguarda una problematica che noi viviamo quasi quotidianamente: la scarsità del servizio taxi. Esso dà la possibilità ai Comuni di aumentare le licenze per quanto riguarda i taxi. Vengono stanziati circa 3 milioni di euro per l'agricoltura e la pesca, in particolare per la cattura del

fino all'ultimo centesimo di quei soldi, perché rappresenteranno il volano della nostra economia e del nostro PIL. E lo abbiamo fatto anche in questo provvedimento, con alcune norme che velocizzano tutta una serie di opere e di infrastrutture ferroviarie, che vengono finanziate e serviranno a rilanciare il nostro Paese

nei piccoli Comuni, negli anni 2023, 2024 e 2025. Molto importante è anche l'articolo 21. Molti Comuni sono in dissesto finanziario e si dà anche a loro la possibilità di riuscire a pagare, con un fondo, i debiti. il contenuto di un decreto che - come detto - sconta un periodo particolare. Siamo, però, ormai entrati nel vivo dell'attività politica e quindi io ritengo che oggi si faccia non un passo indietro, ma rifacciano due passi avanti. Pertanto, ringrazio il Governo per il contributo che ci ha fornito in queste settimane

Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, il decreto *asset*, tra i vari argomenti, ha investito in maniera importante il mondo agricolo, cercando di dare soluzione, in maniera però inadeguata, a due problematiche del comparto: una che attacca la vite,

Più tardi si accetterà questo fatto e più lentamente si potrà risolvere il problema, perché si continuerà a indugiare, aggirando il fulcro della questione senza mai affrontarla con la reale volontà di porre un rimedio efficace. Partiamo dal capitolo delle risorse che - ahimè - è uno dei più amari. Per la peronospora, per ristorare le perdite di migliaia di imprese viticole, il Governo ha pensato, in principio, che fosse addirittura sufficiente solo un milione di euro a livello nazionale. Oggi, in fase emendativa, sono stati aggiunti solo altri sei milioni. respinti tutti i miei emendamenti che chiedevano maggiori risorse. Eppure, l'Italia è storicamente la più grande produttrice di vino in Europa. Solo quest'anno, se le stime verranno confermate, sarà sorpassata purtroppo dalla Francia. questi che convincerebbero anche i non esperti del settore a elargire adeguate risorse per un segmento che è semplicemente trainante non solo per il mondo agricolo italiano, ma per l'intero *made in Italy*. Per il granchio blu, invece, le risorse stanziate sfiorano i tre milioni, ugualmente insufficienti e per di più aggravati dalla raggelante soluzione delle ultime ore proposta dal ministro Lollobrigida, quella di consentire la pesca a strascico entro tre miglia dalla costa. Ma siete davvero sicuri che deturpare l'ecosistema marino sia la soluzione per ridurre la presenza del granchio blu? Le reti a strascico distruggono qualunque cosa incontrino sul fondale: pesci, invertebrati, coralli, alghe, posidonie, lasciando l'*habitat* devastato, privato delle comunità biotiche originarie che si sono formate in tanto tempo e che dunque è indispensabile difendere e preservare. Le reti non sapranno distinguere il granchio blu. Non selezionano il pescato. Dunque, sarà un metodo di distruzione diffuso della ricchezza marina e della biodiversità. L'azione meccanica delle reti, poi, non è solo dannosa per tutte le forme di vita acquatica, ma va anche a intaccare i sedimenti di carbonio, rilasciandoli nell'acqua e innescando un processo di emissione di anidride carbonica. Quindi, per un problema che si pensa di risolvere con un metodo strampalato, se ne creano altri cento di crescente gravità e intensità. I nostri rimedi a entrambe le questioni, peronospora e granchio blu, abbiamo proposto dando una visione prospettica dei fenomeni, affrontandoli con un metodo e non come blanda attenzione Per la peronospora, abbiamo ovviamente chiesto di aumentare le risorse per le aziende colpite, precisando che gli interventi a beneficio delle produzioni viticole devono riguardare l'uva sia da vino che da tavola. Al fine di sostenere la ricostituzione di questa filiera e di contribuire concretamente alla ripresa economica, abbiamo richiesto l'istituzione di un fondo per la rigenerazione della viticoltura. Abbiamo poi pensato a una serie di interventi che potessero affievolire la pressione fiscale sulle imprese agricole colpite dal patogeno in questione, come il contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva in vista del contributo europeo *in de minimis* e il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Coscienti che la peronospora è solo una delle mille facce dell'incidenza antropica sull'ambiente, abbiamo richiesto di dare centralità alla ricerca, attraverso risorse da destinare a studi non solo su questa malattia, ma anche sul rapporto rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole. Questo perché si possa fruire di opportune tecniche che siano adeguatamente attualizzate all'emergenza e al mutato contesto ambientale, giungendo a un concreto contenimento della diffusione del patogeno e aumentando il livello di tolleranza dell'infezione. Per contrastare gli effetti speculativi che stanno imperversando nelle compravendite da uva da vino a uva da tavola, abbiamo proposto un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti proprio le relazioni commerciali tra gli acquirenti e i fornitori. Ciò per garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni e per dare un freno all'inarrestabile volatilità dei prezzi all'origine, che troppo affliggono i nostri produttori agricoli. Ancora, per il granchio blu, abbiamo ritenuto che tra i beneficiari delle misure di sostegno dovessero figurare anche le imprese di lavorazione e di trasformazione circolare dei prodotti dell'acquacoltura e della pesca. Nel dare denaro solo a chi cattura e smaltisce il granchio blu, infatti, il Governo ha perso ancora una volta il *focus* del fenomeno, quello cioè dell'utilizzo e riutilizzo circolare di materiali che differentemente sarebbero classificati in maniera impropria come rifiuti. Rendiamoci conto: il granchio blu diventa un rifiuto. In tal senso numerose aziende, specie di piccole dimensioni, emergenti nel contesto industriale italiano, stanno virtuosamente promuovendo le attività di recupero e di trasformazione di gusci di crostacei in tessuti, impiegati poi in numerosi settori merceologici. È una eventualità anche che - a quanto pare - è stata completamente ignorata. Al momento, infatti, chi vuole regolare la diffusione del granchio blu lo deve fare a suo discapito, quindi a discapito di biosistemi, con costi su costi, in un circolo vizioso senza capo né coda. In ogni caso secondo noi le operazioni di cattura devono essere svolte mediante l'applicazione di metodi di pesca selettiva non impattanti sull'ecosistema e sulla biodiversità locale e attraverso l'utilizzo di tecniche ecologiche tese a ridurre al minimo ogni possibile effetto dannoso. Non parliamo poi delle pratiche di mero smaltimento del granchio blu che, in luogo di usi funzionali, sono solo un ulteriore costo, specie di tipo ambientale. Sempre in un'ottica prospettica e regolatoria abbiamo richiesto che venisse messo nero su bianco un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene e, nello stesso tempo, anche un quadro di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene. Basta ascoltare i centri di ricerca che si occupano dello studio di queste specie per poter agire in modo efficace. Per quanto riguarda il granchio blu, il suo ciclo vitale prevede due fasi: una in acque di transizione (lagune, estuari, porti) e una marina. La maggior parte della loro vita la svolgono nelle acque interne, per poi guadagnare il mare per la riproduzione. È nei canali di comunicazione con il mare, durante i periodi di migrazione, che va catturato, utilizzando le nasse, che sono attrezzi da pesca selettivi. Altro tasto dolente, che non riguarda solo questa trattazione e che sta diventando ormai una pessima consuetudine di questa maggioranza, sta nella presentazione ed approvazione di interventi emendativi che non hanno la benché minima attinenza con il testo in esame. Sto parlando in questo caso degli emendamenti in tema di caccia che distorcono il regolamento sul piombo nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità delle zone umide.

che non si applicherebbe nel caso in cui il soggetto dimostri di detenere le munizioni di piombo - non so - in tasca o nel panino, e quindi non per per andare a caccia ma chissà per cosa. Sarà curioso vedere quindi che spiegazioni verranno date per la detenzione di munizioni di piombo in giro per le aree umide. tratta dunque di un modo subdolo per liberalizzare le attività di caccia, scardinando anche il ruolo di garanzia dell'ISPRA nella definizione dei calendari venatori regionali. Il risultato è che in tutte le zone umide si continueranno a utilizzare le munizioni con il piombo, un vero veleno non solo per la fauna, ma anche per chi consuma poi la cacciagione; ciò nonostante il chiaro divieto disposto a livello comunitario. Le Regioni poi potranno modificare a piacimento la lista delle specie cacciabili - altro abuso - con una grave violazione dei più elementari principi di tutela degli animali. Abbiamo richiesto l'immediato ritiro di questi emendamenti, che minano la credibilità dell'Italia anche nei consessi internazionali, perché proporre delle interpretazioni svianti ed errate delle norme europee significa dare il via a una pioggia di procedure di infrazione, come se non ne avessimo abbastanza. Il Governo, ovviamente, dovrà assumersi la responsabilità di quello che propone e di quello che fa. Come forza di opposizione abbiamo cercato di apportare un concreto contributo: a mia prima firma sono stati approvati tre ordini del giorno e, dunque il nostro grande impegno sembra non sia stato invano, essendo stati recepiti alcuni indirizzi. Per affrontare i problemi bisogna guardare lontano. Non ci si può fermare alla superficie delle cose, senza analizzarle nella loro complessità ed efficacia, per una reale risoluzione nel tempo e non per darne una mera illusione. Presidente, onorevoli colleghi, il cosiddetto decreto *asset* racchiude una serie variegata di misure che riguardano ambiti anche lontani tra loro per i quali è richiesto con urgenza il nostro intervento. misure e ambiti che toccano, infatti, direttamente o indirettamente, le tasche degli italiani, le loro attività economiche, i loro spostamenti e le infrastrutture connesse, e quindi incidono pesantemente sulla loro vita personale quotidiana. Verso di loro l'attenzione di questo Governo è stata ed è sempre massima.

criticata, il Governo si preoccupa di garantire la massima trasparenza dei prezzi praticati sui voli nazionali con una particolare attenzione a una parte dell'Italia troppo spesso non considerata, ovvero le isole, e io, da siciliano, ne sono testimone. Per farlo si rafforzano i poteri dell'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, che valuterà in tal modo le tariffe. Si tratta di un provvedimento importantissimo non solo per i viaggiatori ma anche per la stessa economia del Paese. Il trasporto aereo è uno strumento fondamentale per lo sviluppo degli affari e, se un viaggio costa troppo o addirittura diventa proibitivo e non conveniente, rappresenterà un danno, una gravissima perdita di opportunità di crescita e sviluppo per i territori interessati. Ecco perché tale previsione va condivisa da tutti. Questo è lo spirito che muove, in generale, l'azione di questa maggioranza e del Governo. Un altro esempio è quello del trasporto taxi. Il nostro Ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, da tempo interloquisce con la categoria dei tassisti che gli hanno sottoposto le giuste rivendicazioni per i costi sostenuti per le licenze e soprattutto, oggi, per i costi del carburante e della manutenzione delle auto. Sappiamo anche, però, quanto attualmente il servizio sia insufficiente, soprattutto nelle grandi città, con enormi disagi per la cittadinanza e purtroppo anche con un danno di immagine per l'Italia agli occhi dei turisti, che spesso non riescono a trovare mezzi per spostarsi in maniera veloce. Finalmente si fa attenzione anche alle piccole comunità. L'articolo 19 istituisce presso il MIT un fondo di investimenti stradali nei piccoli Comuni con una dotazione di 50 milioni di euro per le annualità 2023-2024 e 2025 che potranno usare per mettere in sicurezza manutenere strade, ponti e viadotti. Ricordo anche l'anticipo di liquidità per i Comuni in dissesto, che purtroppo sappiamo essere sempre di più nel nostro Paese. Cito altre misure, come ad esempio come ad esempio le norme per consentire la piena e rapida operatività della neonata - o rinata - Stretto di Messina SpA, la concessionaria per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, e la Calabria, al fine di realizzare nei termini previsti tutte le complesse attività funzionali alla realizzazione dell'opera. Aspettiamo con ansia anche il disegno di legge di bilancio per inserire i primi fondi e zittire un po' di uccellacci del malaugurio. Ricordo la cassa integrazione straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico o per i dipendenti dell'Alitalia, viene prevista una proroga dell'integrazione salariale fino all'ottobre 2024, in modo da accompagnare i processi di ricollocazione. Per il settore della pesca - come è stato più volte richiamato - è stato un contributo per fronteggiare la diffusione ormai invasiva del granchio blu che sta provocando gravi danni nel settore ittico e all'acquacoltura. E ancora, citerei il fondo istituito presso il MEF per gli interventi di bonifica, di ricostruzione e di messa in sicurezza dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali: più di 100 milioni per il 2025 e più di 100 per il 2026. Ci sono, inoltre, interventi per le aziende agricole che hanno subito danni alle produzioni vitivinicole non coperti da risarcimenti assicurativi; c'è il fondo da 15 milioni di euro per ristorare viaggiatori e operatori del settore turistico colpiti purtroppo quest'estate dagli incendi sia in Sicilia che in Sardegna; un incremento a quasi 150 milioni di euro per il 2023 del contributo per la ricostruzione dei territori colpiti dalle alluvioni (Emilia-Romagna, Toscana, Marche); cito il rafforzamento del contrasto della delocalizzazione con la previsione che le grandi imprese che hanno beneficiato degli aiuti di Stato non possono delocalizzare la produzione prima di dieci anni anziché cinque.

come hanno già ricordato alcuni colleghi, stiamo affrontando in quest'Aula un provvedimento che nulla ha a che vedere con il nome che gli era stato assegnato, ossia decreto *asset*. Credo sia inutile ricordare che i provvedimenti d'urgenza devono recare misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di applicazione immediata. Come è evidente a tutti noi, questo è solo un vero e proprio provvedimento *omnibus*, contenente le più svariate disposizioni che nel corso della sua conversione ha subito interventi, tanto da parte del Governo quanto da parte della maggioranza, che lo hanno ulteriormente snaturato. Qualcuno avrebbe davvero il coraggio di argomentare che non sia così? Abbiamo affrontato tematiche che hanno spaziato dall'estensione dei poteri speciali - la *golden power* - per i settori ad alta tecnologia al contenimento del granchio blu. I provvedimenti per l'emergenza del disastro alluvionale in Emilia-Romagna hanno avuto meno spazio della deroga ai pallini al piombo per i cacciatori. Invece di approfondire le politiche industriali per il comparto strategico dei *microchip*, la maggioranza ha tentato fino all'ultimo di tenere l'attenzione sugli allevamenti per i cavalli da corsa. Un provvedimento così disomogeneo e con caratteri talmente diversificati avrebbe avuto bisogno almeno di una presenza costante dell'intero Governo, di tutti i Ministeri, di una approfondita discussione nelle Commissioni competenti. Invece, nonostante la correttezza istituzionale che riconosciamo ai due Presidenti di Commissione, il Governo ha portato ancora una volta il Parlamento a essere spettatore, costringendo all'esame di oltre 500 emendamenti - lo ha ricordato il relatore - in poco meno di due giornate, con continui rinvii in attesa dei pareri dei tanti diversi Ministeri coinvolti e sfruttando il provvedimento per inserire ulteriori norme che nulla avevano a che vedere con le finalità dello stesso. Altri colleghi affronteranno le tematiche di così grande valenza che il decreto si riprometteva di risolvere e invece ha lasciato irrisolte. Io vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea su due di particolare rilevanza. rilevanza. Mentre la maggioranza di Governo litigava solo di extraprofitti alle banche, prima annunciati e poi nella pratica ritirati su imposizione di Forza Italia, il Paese attendeva risposte su questioni dirimenti come la ricostruzione in Emilia-Romagna e la risoluzione dei crediti incagliati che stanno bloccando opere in tutto il Sul tema ricostruzione *post* alluvione in Emilia-Romagna, assistiamo al totale fallimento delle scelte iniziali che il Governo ha compiuto: propaganda, dichiarazioni di 4,5 miliardi di euro a disposizione per la ricostruzione. Nella realtà, tutta la frammentazione introdotta dai diversi Ministri con misure individuali dei singoli Ministeri fatte a *spot* sta determinando l'impossibilità dell'utilizzo anche delle poche, scarse risorse assegnate, per cui oggi siamo ancora alla metà delle risorse disponibili rispetto al fabbisogno necessario per ricostruire strade, per rimettere in sicurezza tutta la montagna e l'Appennino. Ma, soprattutto, di fatto queste sono le prime risorse risorse a disposizione del commissario per indennizzare famiglie e imprese; risorse che sono abbondantemente lontane dal miliardo di euro quantificato. Siamo quindi in presenza di un tradimento delle promesse che la presidente Meloni e diversi Ministri, nelle varie sfilate elettorali che hanno compiuto subito dopo l'alluvione, avevano garantito, promettendo di indennizzare i danni non solo non sono stati ancora indennizzati, ma hanno compromesso anche la vita di molte aziende. Le imprese, infatti, rischiano di non avere le condizioni - sul versante dei loro bilanci - per poter garantire una ripartenza ordinata delle loro attività,

lasciando sconnesse tante realtà. Siamo in grande ritardo per colpa di un progetto sbagliato e delle scelte sbagliate di questo Governo, che ha fallito e sembra non volersi rendere conto dei propri errori. *(Applausi)*. Anche sul superbonus imprenditori e famiglie sono stati ancora una volta mortificati dal Governo che, insieme alla maggioranza, ha bocciato tutti gli emendamenti in materia. A nulla sono serviti gli appelli forti non solo di migliaia di cittadini e lavoratori preoccupati, ma anche di rappresentanti delle tante categorie economiche che da mesi denunciano i rischi di questa inerzia. Con un nostro emendamento avevamo richiesto la necessaria proroga al 31 dicembre 2024 per i lavori nei condomini, ma tale proposta è stata bocciata; medesima sorte addirittura per gli emendamenti della maggioranza che prevedevano una proroga almeno al 30 giugno 2024. Tutto questo mentre la vera questione, quella dei crediti incagliati, mette in ginocchio esodati del superbonus e imprenditori onesti che si sono fidati dello Stato, ma sono ormai relegati sempre più nel totale disinteresse dell'Esecutivo. Governo e maggioranza sono stati sordi davanti alle difficoltà che mettono in ginocchio famiglie e imprese. famiglie e imprese. Tuttavia, non hanno lesinato risorse per finanziare la società Ponte sullo Stretto di Messina, per dare incarichi commissariali con nuovi oneri per le finanze pubbliche secondo una logica spartitoria dei partiti di maggioranza. Avevate mai visto creare commissari di Governo con emendamenti parlamentari, oppure rischiare nuove infrazioni comunitarie, ricorrendo a finanze pubbliche per derogare all'uso dei pallini al piombo? La verità è che, di fronte alle tante mancate promesse di questa maggioranza, in vista di una legge di bilancio in cui i partiti di maggioranza hanno compreso che non troveranno risorse per tante promesse elettorali, è stato usato il decreto-legge in esame per contendersi i fondi disponibili, invece che per affrontare seriamente le tante urgenze del nostro Paese. D'altra parte, abbiamo e avete avuto difficoltà anche a dare un nome a questo zibaldone; magari sforzandoci potremo paragonarlo alla pioggia: norme, provvedimenti, risorse a pioggia senza un'idea, una visione, una direzione, una qualche intelligenza razionale. Purtroppo, alla fine resterà una pioggia destinata a non trovare un contenitore e a evaporare presto, lasciando troppe domande senza risposte e troppe aspettative delle italiane e degli italiani dolorosamente tradite. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n.

Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame oggi è solo l'ultimo importante tassello che negli ultimi mesi Governo e Parlamento hanno realizzato insieme in tema di imprese, semplificazione, crescita e investimenti strategici. In soli dieci mesi di buon governo del centrodestra, come provato da ogni dato economico, diverse sono state le misure approvate per favorire la crescita delle imprese e la competitività del comparto industriale italiano, lungo quel percorso già tracciato dal presidente Meloni e che riteniamo possa assicurare pieno sviluppo al Paese, nell'ottica di un rilancio nazionale e della competitività delle nostre imprese italiane, di quegli *asset*, appunto, che sono strategici per far fare gol al Paese e che questo decreto intende promuovere, tutelare e rafforzare. In ragione di questo interesse nazionale, l'articolato decreto-legge in esame mira a varare importanti misure in favore di settori fondamentali della nostra economia: dal settore dei trasporti a quello dell'agricoltura e pesca, dal settore turistico-ricettivo a quello energetico, dalla velocizzazione dei cantieri previsti dal PNRR alla competitività delle imprese sui mercati internazionali. Penso in particolare alle norme per far fronte alle carenze del sistema di trasporto pubblico a mezzo taxi: le file interminabili di turisti e cittadini comuni ai varchi delle stazioni e degli aeroporti, ad esempio nelle grandi città come Roma e Milano, sono inaccettabili e non sono degne di un Paese civile come il nostro, che fa del turismo il proprio biglietto da visita. disperazione dei turisti che perdono aerei e treni per assenza di mezzi di trasporto pubblici è un deterrente per un Paese la cui economia può gemmare quasi esclusivamente sul turismo. Penso in particolare al tema dell'accesso al credito per le imprese o anche ai problemi legati ai ritardati pagamenti dei lavori eseguiti in favore della pubblica amministrazione, oppure ai tanti crediti fiscali ancora incagliati a causa di scellerati *bonus* distribuiti a pioggia (uno per tutti, il superbonus, voluto dai precedenti Governi di centrosinistra), che ora influiscono forse negativamente negativamente sulla manovra finanziaria che il Governo si appresta a varare, e che quei Governi hanno varato senza pensare a quello che avrebbero successivamente causato al bilancio dello Stato e soprattutto al futuro delle nostre generazioni. Penso anche all'eccessiva pressione fiscale che grava ancora su quelle imprese che vogliono investire in particolare in innovazione, specie quella digitale, un settore che merita di essere accelerato e tutelato, perché *start up* e innovazione tecnologica rappresentano oggi un *asset* strategico fondamentale e al tempo stesso un importante fetta del nostro PIL nazionale. D'altronde, sono i dati e le statistiche che lo certificavano, come dirò più innanzi. Per essere seri e concreti, però, dobbiamo garantire loro un quadro di maggiori certezze che favorisca e non certo penalizzi gli imprenditori, proseguendo nella scia di sburocratizzazione, eliminando lacci e lacciuoli che da troppo tempo attanagliano le nostre imprese. Presidente, nel provvedimento che stiamo esaminando abbiamo voluto ricordare anche un altro settore strategico per la nostra economia: mi riferisco al settore turistico e in particolare al tema delle concessioni demaniali. Gli imprenditori turistico-balneari meritano la giusta attenzione, soprattutto alla luce delle recenti pronunce del Consiglio di Stato, tali da complicare non poco il tema del rinnovo delle concessioni. In tale ottica, noi non ci siamo mai sottratti al confronto, facendoci parte attive e proattiva di questa maggioranza. pertanto il Governo per aver dimostrato sensibilità e ascolto verso un tema così delicato, posto da subito alla sua attenzione: il tema dei canoni per le concessioni. Si poteva fare però di più in merito alle concessioni rilasciate a chi intende usare il patrimonio pubblico demaniale marittimo per fare impresa senza scopo di lucro e senza sfruttare economicamente le aree demaniali rilasciate in concessione *(Applausi)*: un primo importante punto fermo, un solido riconoscimento a chi della categoria fa impresa etica, lasciando che le nostre coste e il nostro mare possano davvero essere patrimonio di tutti e gratificare il territorio. Da ultimo, signor Presidente, ma non per questo meno importante, voglio richiamare l'attenzione del Governo e dell'Assemblea verso un settore parimenti

Per quanto riguarda il raffronto con altri Paesi, basti pensare che nel 2022, un anno *record*, in Italia sono stati investiti circa 1,8 miliardi sulle *start up* e le imprese innovative; un dato che invece viene triplicato, se non moltiplicato, in altre realtà. Nonostante gli alti e bassi, l'ecosistema italiano dell'innovazione sta attraversando una fase di crescita. Ci sono le basi per essere il prossimo potenziale centro di attrazione per molti operatori internazionali, come dimostrato da una crescita del 48 per cento del mercato del nostro Paese

Ci auguriamo quindi che, come segno di attenzione verso un settore così strategico per la crescita, per l'internazionalizzazione e la competitività dell'Italia nel mondo, ben presto possano essere varate misure che sappiano tutelarne e promuovere gli interessi. Ricordo che ogni singolo euro investito in economia dell'innovazione rappresenta un euro in più restituito alle future generazioni. Mi avvio a concludere. La nostra visione riteniamo sia quella di realizzare un contesto più competitivo per le imprese e più attrattivo nei confronti di nuovi capitali e investimenti, nonché di salvaguardare gli interessi strategici nazionali, in coerenza con gli interventi interventi di interesse comune per le industrie italiane ed europea. In tal senso, abbiamo ben chiara la strategia da seguire, come ha detto il *premier* Meloni da quando ha assunto la responsabilità di Governo. Il monito che credo sia il più importante e che ciascuno di noi dovrebbe rammentare è solo uno: tornare a crescere per far tornare grande l'Italia. Continueremo Siamo convinti che il Paese o, per meglio dire, la squadra Italia saprà reagire e ce la farà, se ognuno,

Presidente, ci troviamo ancora una volta, anzi per l'ennesima volta, davanti a un decreto-legge che approvate con la fiducia, un decreto peraltro che avrebbe dovuto trattare urgenti interventi strategici per lo sviluppo del Paese. infatti chiamato inizialmente decreto *asset*, ma strada facendo - come è stato riportato e detto da molti colleghi - è diventato un vero e proprio decreto *omnibus*, con al suo interno norme di tutti i tipi e del tutto eterogenee, che riguardano argomenti diversissimi tra di loro, alcuni dei quali sono effettivamente urgenti, mentre tanti altri sono di ordinaria amministrazione, sui quali evidentemente il Parlamento avrebbe dovuto esprimersi con il procedimento ordinario. Si passa dalle tariffe aeree ai granchi blu, dal trasporto pubblico locale alla ricostruzione post-alluvione, dalla micro-elettrica alla pesca, dall'Alitalia alla TIM. Si parla di caccia, si parla di foreste; verrebbe davvero da domandarsi cosa c'entrino, per esempio, i pallini di piombo, di cui ha parlato poc'anzi la nostra senatrice Floridia, con l'*asset* strategico del Paese, tanto per dirne una. Mi sembra - mi dispiace dirlo - che siano ancora una volta cadute del tutto inascoltate le sagge parole e le sagge raccomandazioni dello stesso Presidente della Repubblica, che tante volte, volte, anche negli ultimi mesi, ha invitato a non inserire norme palesemente eterogenee rispetto all'oggetto e alla finalità dei provvedimenti d'urgenza. Ma è chiaro che il Governo ha scelto la strada di andare avanti, ignorando tutto e tutti, e presenta per l'appunto quello che noi consideriamo un vero e proprio obbrobrio. Nel merito delle misure, la prima cosa che vorrei evidenziare è che, anche su quelle poche scelte un po' più coraggiose che per una volta il Governo aveva cercato di mettere all'attenzione, si è però poi scelto di tornare indietro. Ciò è successo attraverso una serie di emendamenti presentati in Commissione;

con un risultato finale che ci sembra del tutto deludente. Ancora una volta, una vera e propria montagna che partorisce il topolino. Mi riferisco in particolare, Presidente, agli articoli 1 e 2, sulle tariffe praticate sui voli nazionali, in particolare sulla decisione di fissare una soglia massima alle tariffe, per evitare che si ripresenti di nuovo il problema che si è verificato questa estate, cioè tariffe gonfiate a dismisura anche su tratte di continuità territoriale (penso alla Sicilia e alla Sardegna in particolare), con la conseguente insopportabile compressione del diritto di movimento delle persone, particolarmente grave, peraltro, quando si tratta di isolani a cui viene imposto il pagamento di cifre esorbitanti per poter tornare a casa o per poter ripartire da casa. Avete deciso di fissare una soglia massima agli aumenti delle tariffe, ma, di fronte alle lamentele delle compagnie aeree, avete fatto clamorosamente dietrofront, dimostrando davvero pressappochismo e anche una certa improvvisazione fatemela definire così - mentre invece io credo - come ho sempre detto in tutti questi mesi - che il Paese avrebbe più che mai hai bisogno di grande competenza e di grande serietà. Stessa cosa, se possibile ancora più grave, per quanto riguarda la cosiddetta norma sugli extraprofitti delle banche. L'avevate presentata inizialmente come una misura di equità sociale. Sono da ricordare oggi le parole del ministro Salvini di qualche settimana fa sui giornali, era la convinzione che il prelievo sui maximargini delle banche che hanno guadagnato decine di miliardi in questo periodo fosse la strada giusta per aiutare lavoratori, famiglie ed imprese. Parole giuste: peccato, però, che poi siano state totalmente disattese da quello che è successo nel corso delle settimane successive. Anche su questo, totale e clamoroso dietrofront del Governo. Peraltro, il danno e la beffa, perché c'è stato, nel frattempo, anche il crollo di Piazza Affari, con le inevitabili polemiche della stampa internazionale, che ovviamente ha considerato goffo e caotico questo modo di fare. Ancora una volta, anche in questo caso mi pare abbastanza evidente come si sia vista tutta la debolezza di una coalizione purtroppo non sufficientemente capace, dal mio punto di vista, di guidare autorevolmente il Paese. Sempre la solita logica: grande forza con i fragili e invece grande debolezza con i forti. Tanto per citare un altro esempio, ma davvero si potrebbe andare avanti per ore in questa disamina, pensate alla vicenda TIM e al fatto che siano rimaste inascoltate le istanze di chi chiedeva che un così ingente investimento di risorse pubbliche venisse vincolato a precisa garanzia di stabilità sui posti di lavoro in gioco, che peraltro sono molte migliaia. Invece, il timore è che fra qualche mese dovremo affrontare le conseguenze di spregiudicate delocalizzazioni all'estero di lavoratori in esubero, gestiti, come sempre, come numeri e non come persone in carne ed ossa: esattamente come sta accadendo in queste ore ad i lavoratori ex Alitalia. Problemi, insomma, che riguarderanno interi settori ed interi comparti; sembra, però, che davvero i destini di queste persone interessino poco. Sono state peraltro bocciate proposte emendative bocciate proposte emendative di puro buonsenso: una per tutte, quella tesa ad evitare una vera e propria stortura del nostro ordinamento, che prevede l'obbligo di restituzione degli ammortizzatori sociali fruiti da lavoratori reintegrati giudizialmente anche dopo diversi anni trascorsi dal licenziamento illegittimo. È una questione che peraltro riguarda moltissimi lavoratori, che hanno atteso magari per anni una sentenza che, per l'appunto, cancellasse l'illegittimo licenziamento e che però prevede, come indennizzo, una somma equivalente a un solo anno di retribuzione. Sarebbe stato assolutamente giusto intervenire su questo, ma non è stato fatto. Avete rigettato istanze del tutto meritevoli, come questa di cui ho appena detto, per accoglierne altre discutibili. Mi riferisco, in questo caso, agli emendamenti che avete approvato in tema di caccia. Anche qui, davvero si fa fatica a comprendere quale sia stata la traccia che tenesse insieme questi argomenti diversi. Anche in questo caso, avete stravolto totalmente l'equilibrio della competenza tra Stato e Regioni. Evidentemente è un tema, quello della competenza Stato-Regione, che vi appassiona molto, perché voi siete gli stessi che, in queste

avete svilito il ruolo dell'ISPRA, in sostanza annullando il valore del parere, che può essere superato con una cosiddetta motivazione adeguata. Anche in questo caso,

di regalare ai dirigenti della società Ponte dello Stretto di Messina la soppressione del tetto dei 240.000 euro agli stipendi degli amministratori, titolari e componenti degli organi di controllo.

da una totale diseguaglianza, dalla grande evasione che purtroppo conosciamo bene, dall'immunità penale e dalle questioni di cui abbiamo discusso molte volte. Esattamente mentre tagliate questo tetto è, in qualche modo, fate questi regali milionari, abolite però il reddito di cittadinanza e lo trasformate in una vera e propria elemosina di Stato. Continuate con questo racconto sloganistico secondo il quale ci sarebbero i giovani seduti sul divano che non vogliono lavorare, mentre tutti sappiamo che il reddito di cittadinanza era anche e soprattutto uno strumento per evitare che quei giovani, quelle ragazze e quei ragazzi, fossero fossero sfruttati sul lavoro, visto che molto spesso vengono loro proposti 3 o 4 euro all'ora per andare a lavorare. Ecco, francamente, dinanzi a questa clamorosa sperequazione, mi sembra davvero che ci sia ben poco da aggiungere.

profondamente contrario del Gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo,

passata legislatura l'opposizione, soprattutto Fratelli d'Italia, ci accusava spesso di mettere la fiducia perché non eravamo coesi su nulla,

ai danni dei cittadini; guardiamo il caro volo. Tra l'altro, l'incontro con le compagnie aeree è stato organizzato dal ministro Urso - non ho capito perché non dal ministro Salvini - alla fine dell'estate, quando cioè ormai il caro voli sulle Nonostante questo, fate anche una norma, in questo caso, completamente sbagliata, solamente di chi vi parla, ma dell'Unione europea, che comincia a sollecitare un passo indietro rispetto alla norma che prevedeva un tetto massimo al prezzo dei voli, oltre ovviamente alla protesta di tutte le compagnie aeree e, di fatto, al blocco operato da Ryanair da Ryanair dei viaggi dalle isole al continente, con un danno ulteriore ai cittadini italiani. Avete fatto allora marcia indietro, ma non soltanto in questo caso. Avete fatto marcia indietro praticamente un po' su tutto, in particolare sulla norma sugli extraprofitti bancari. Chi vi parla pensa che quella norma fosse una grande sciocchezza. L'articolo 47 della Costituzione dice che

la sorpresa dei mercati finanziari all'annuncio di una tassa, scritta tra l'altro male, tant'è vero che avete dovuto fare marcia indietro anche su questo argomento,

ABI, Banca d'Italia e delle maggiori banche, chiedendo un contributo di solidarietà? Avreste avuto forse meno titoli sui giornali come "il Governo bacchetta le banche" e magari meno *like*, ma avreste avuto le risorse che così intanto non avete *(Applausi)*, la norma che avete riscritto, di fatto, non vi farà avere i 10 miliardi che avevate preventivato su quel capitolo. Com'è stato detto da molti

piccole nicchie di interesse che non sono però l'*asset* strategico del nostro Paese. Un anno fa - è vero che bisogna ricordare quello che è successo - un Governo è caduto sui tassisti e sulle licenze balneari. Dopo un anno, il problema dei taxi non è stato risolto, neanche con questo provvedimento, perché di fatto rimane tutto inalterato, di fatto i cittadini continueranno a fare la coda e il taxi sarà una chimera (perché non abbiamo risolto neanche il problema degli NCC), quindi su quell'argomento avete deciso di abdicare e di non decidere, che è meglio, perché ovviamente avere contro una *lobby* importante come quella dei taxi fa male. Certamente bisognerebbe avere il coraggio di andare in piazza a confrontarsi con persone che non sarebbero sicuramente felici di avere una concorrenza più ampia, ma magari i cittadini, che in questo momento fanno code interminabili e si trovano un disservizio così elevato nel nostro Paese, avrebbero sommessamente ringraziato il Governo per aver pensato a loro. Insomma, il decreto al nostro esame non risolve i problemi degli italiani, dà mance più o meno piccole ad alcuni portatori di interessi particolari, che non sono la struttura ossea dell'economia del nostro Paese, e poi però

perché sono limitata io - la strategia per TIM, la sua modernizzazione e la salvaguardia dei posti di lavoro, ma anche per l'incentivazione di quella che dovrebbe essere finalmente la rete unica, per poi arrivare al 5G. molto rumore per nulla e penso che ve ne siate accorti anche voi, perché ad un certo punto non arrivavano neanche i pareri sulle riformulazioni del Governo. Noi non abbiamo dovuto fare, come opposizione, alcun ostruzionismo. Ci avete pensato voi. Avete sconvocato le Commissioni della scorsa settimana perché non eravate pronti. Questa è una settimana particolare, che è iniziata ovviamente con il lutto nazionale per rispetto del presidente Napolitano - e ci mancherebbe - ma mercoledì e giovedì sono giorni che hanno visto la fatica di questa maggioranza per arrivare alla conclusione del provvedimento in esame, perché forse anche voi, cammin facendo, avete perso le parole di entusiasmo che avevate pronunciato non appena pubblicato decreto-legge, rendendovi conto che alla fine non avete portato a casa nulla per l'economia del Paese. Sapete che cosa lo certifica, visto che dai vostri banchi ogni volta si parla delle misure e degli indici macroeconomici che rendono solido il nostro Paese? I tassi di interesse e la differenza che c'è tra i nostri tassi di interesse e quelli tedeschi e quella che c'è tra i tassi della Grecia e quelli tedeschi: stiamo peggiorando. Siamo stati superati in meglio dalla Grecia: ma come, non era uno spauracchio non finire come la Grecia? Bene, siamo finiti molto peggio: grazie di questo regalo!

Lo fa attraverso un ampio e ragionato articolato, che prevede misure mirate su alcuni aspetti critici della nostra economia, innanzitutto attraverso norme che incentivano gli investimenti delle imprese e l'iniziativa dei privati, ma anche attraverso alcuni divieti, come quello di delocalizzare da parte di imprese che abbiano ottenuto aiuti pubblici. Allo stesso tempo, contiene norme a tutela dei consumatori e interviene per sostenere progetti di ricerca e sviluppo, attraverso i quali si guarda in maniera prospettica allo sviluppo della nostra economia.

anche se pochi lo sanno - è protagonista: basti pensare che proprio nel mio Piemonte, a Volpiano, si trova una delle tre aziende *leader* mondiali della verifica automatizzata dei *microchip*. L'esame in Commissione ha visto anche diverse modifiche, mirate a correggere quella che nel testo iniziale lo stesso vice *premier* Tajani aveva evidenziato come criticità. Mi riferisco alla tassazione dei cosiddetti extraprofitti delle banche. Se da un lato le banche si sono trovate, in un momento di rialzo dei tassi di interesse da parte delle banche centrali di tutto il mondo, ad avere un margine di interesse maggiore e hanno guadagnato col salire dei tassi, non hanno però remunerato proporzionalmente i risparmi degli italiani. Dall'altro lato, però, il modo in cui inizialmente si era provveduto a tassare questo maggior profitto presentava molti rischi per i correntisti, soprattutto quelli delle piccole banche. Le richieste di Forza Italia hanno portato a un proficuo confronto all'interno del Governo e del Parlamento, producendo una soluzione condivisa da tutta la maggioranza. È stata quindi modificata la base imponibile dell'imposta, in quanto ora viene applicata sull'attivo medio ponderato, che porta all'esclusione dei titoli di Stato dalla tassazione, per evitare di disincentivarne l'acquisto da parte del sistema bancario italiano in considerazione della sua capacità di assorbire quote rilevanti del debito pubblico. Inoltre, viene concessa a ogni istituto di credito la possibilità di scegliere tra versare l'imposta oppure rafforzare il proprio capitale, mettendo a patrimonio due volte e mezzo il valore dell'imposta dovuta. Questo consentirà soprattutto alle piccole banche di patrimonializzare l'imposta, rafforzando la solidità dell'istituto stesso, mettendo quindi in sicurezza i correntisti e consentendo una maggiore concessione di credito sia ai privati sia alle imprese. Inoltre, come aveva rilevato la stessa BCE, maggiori riserve consentiranno di affrontare in sicurezza eventuali esercizi in perdita nel futuro. Questo vuol dire che in Italia non ci saranno più questioni come quella del Monte dei Paschi di Siena o, per pensare a un dramma mondiale, della Lehman Brothers. Invece, le banche più solide e maggiormente orientate alla distribuzione di utili ai propri azionisti faranno le proprie scelte: se verseranno l'imposta, contribuiranno a finanziare gli scopi previsti dal decreto-legge, che non vengono meno, come l'aiuto alle famiglie che stipulano mutui per l'acquisto della prima casa o il rifinanziamento del Fondo per le piccole e medie imprese. Infine, è stato previsto che le banche non potranno rivalersi

Parliamo di territori che scontano già una discontinuità territoriale che non può essere aggravata da costi per biglietti che a volte crescono in maniera immotivata. Sui prezzi dei voli, che non possono essere regolati da algoritmi, avrà potere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato: si tratta di poteri ampi e articolati che possono verificare il funzionamento degli algoritmi, al fine di evitare il crearsi di pratiche concordate o di posizioni dominanti. Anche su questo intervento la tutela del consumatore è stata l'obiettivo principale dell'azione della maggioranza di Governo. Una ulteriore questione sulla quale si è fatta molta speculazione politica sulle spalle di gente che certamente non lo meritava riguarda i sostegni alle zone alluvionate del maggio di quest'anno. Anche in questo ambito il Governo si è mosso con grande trasparenza e senza strumentalizzazioni, innanzitutto nominando un commissario che gode di una stima e di un apprezzamento molto ampi, il generale Figliuolo, e ora con il decreto-legge in esame il Governo interviene rifinanziando le risorse destinate ai contributi economici per gli eventi di ricostruzione privata nei territori dell'Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche. le risorse ci sono e vengono assegnate a chi ne ha diritto. Mi sono soffermato su alcune modifiche proposte al testo iniziale del decreto-legge, che contiene molte altre misure, soprattutto di sostegno al nostro vasto tessuto di imprese e al mondo del lavoro. Infine, durante l'esame in Commissione sono stati accolti diversi emendamenti di Forza Italia volti a migliorare il testo del provvedimento: come sempre, l'ascolto delle categorie e del Paese reale ha avuto un ruolo importante nella nostra attività emendativa.

e la maggioranza di centrodestra dimostra per l'ennesima volta di essere in grado di garantire il rispetto della volontà di noi rappresentanti del popolo: abbiamo esaminato uno per uno 550 emendamenti e ne sono stati approvati molti, anche dell'opposizione. Abbiamo inoltre dimostrato che questa maggioranza riesce a fare sintesi anche delle diverse sensibilità delle forze che la compongono. Per questi motivi, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi ci ritroviamo ancora una volta a discutere delle scelte a metà di un Esecutivo che pare procedere per tentativi: esame, così come gli altri, sostanzialmente è infatti andato sgonfiandosi in significato e contenuti fin dai primi giorni. A pensarci bene, è eccessivo anche parlare di scelte, fatto non far nulla è la conseguenza di decisioni non prese, a meno che non abbiate deciso che sia proprio questa la vostra scelta, la vostra linea politica.

narrando una favola a cui ormai solo voi credete e in ogni caso di questa fantomatica corsa si percepisce esclusivamente il vostro affanno. È di favole che avete riempito la vostra politica e la vostra campagna elettorale: oggi sembrate delle mummie costrette nelle bende della vostra arroganza e delle promesse impossibili da realizzare. *(Applausi)*. che avete messo gli occhi sul Museo egizio di Torino: forse siete alla ricerca di un comodo sarcofago in cui nascondervi dalla vergogna, in attesa che passi la tempesta.

a quest'Assemblea e all'intero popolo manca ancora la percezione, non si è ancora compreso se siete partiti e e che cosa avete fatto. Ah no, perdonatemi, dimenticavo l'urgenza e la necessità della legge sulla carne sintetica, che è arrivata nel momento in cui il divieto era già vigente. *(Applausi)*. Andiamo nel merito del provvedimento che ci apprestiamo a votare. Prendiamo ad esempio l'articolo in cui avete sostanzialmente spogliato l'Autorità di regolazione dei trasporti di funzioni ad essa riconosciute da leggi e sentenze, funzioni insite nel ruolo stesso dell'Autorità; avete escluso dai principi di equità e non discriminazione un'unica categoria, quella degli autotrasportatori di merci, e avete deciso di tirare dritto per questa strada, anche davanti a una serie di perplessità che la stessa Autorità di regolazione dei trasporti ha sollevato durante il corso delle audizioni nelle Commissioni Commissioni riunite, andando incontro, con ogni probabilità, a dubbi di tenuta costituzionale della normativa da voi inserita e sotto il profilo della disparità di trattamento tra gli operatori economici. Tutto questo

Sulla questione delle tariffe dei voli, il ministro Urso, che per la verità non è nuovo all'improvvisazione, è stato costretto a una clamorosa marcia indietro: lo dico ai colleghi di maggioranza che negano questa evidenza. C'è stata una clamorosa marcia indietro, perché ricordiamo quando il Ministro settimane fa tuonava che non fatti ricattare da Ryanair. Sappiamo bene quale sia stato nei fatti il risultato di cotanta fermezza: è stato presentato un emendamento governativo che ha riscritto l'articolo in questione, che in buona sostanza si è limitato a rafforzare i poteri dell'Antitrust. In sintesi: un atterraggio morbido, da applausi per le compagnie e a discapito degli utenti. *(Applausi)*. L'algoritmo usato dalla maggioranza e dal Governo è sempre lo stesso, al pari del risultato, chiaramente. La formula prevede un annuncio altisonante a reti unificate contro questo o quel sistema che deve essere distrutto e successivamente lo si aiuta a prosperare. Vogliamo parlare degli extraprofitti delle banche? È arrivato il momento La norma è stata annunciata come una vera e propria rivoluzione. Chi si scorda di Giorgia Meloni pronta ad affermare di essersi presa la responsabilità di averla fatta inserire nel testo senza condividerla con il Governo? Insomma, una di quelle operazioni da "io ci metto la faccia". Anche noi del MoVimento 5 Stelle, con gran stupore, devo dire, avevamo accolto con un certo entusiasmo questa decisione presa dal Governo, visto che sono mesi che chiediamo di intervenire sugli extraprofitti (non solo delle banche, perché noi parliamo anche di quelli di di assicurazioni, case farmaceutiche, imprese energetiche e industria delle armi). *(Applausi)*. Ebbene, tanto rumore per nulla, a conferma di quanto vi dicevo poc'anzi. Avete riscritto la norma per ben tre volte per placare le tensioni della maggioranza,

sarà dato dalla differenza tra l'esercizio del 2021 e quello del 2023, che è ancora in corso, quindi l'entrata non è quantificabile. La genialata sta però nell'aver garantito alle banche la possibilità di evitare l'imposta, versando una somma per rafforzare il proprio patrimonio. Il risultato? Gettito impossibile da prevedere. Secondo voi - sono curiosa di capire - quale banca deciderà di pagare una tassa invece di autofinanziarsi? Mi aspetto una risposta negli interventi che seguiranno. Complimenti, quindi, anche per questa bellissima trovata. Viene da pensare che lo abbiate fatto apposta, perché l'alternativa è quella di ritenervi assolutamente incapaci. Noi abbiamo provato a cambiare questa norma, al pari di altre; lo abbiamo fatto con diversi emendamenti e il senatore Turco lo sa bene; lo ringrazio per il suo contributo, ma purtroppo non siamo riusciti a cambiare questa norma. Anzi, permettetemi di ringraziare tutti i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che hanno lavorato con il loro impegno e con una decisa volontà

un grosso favore alle banche. *(Applausi)*. In Commissione avete respinto tutti gli emendamenti che abbiamo proposto sul superbonus; anzi no, avete respinto anche i vostri. Da un anno stiamo assistendo ad uno spettacolo indecoroso fatto di attori e comparse che dicono che andrà tutto bene, perché loro amano metterci la faccia. Ma quelle che vediamo sono solo delle maschere che sussurrano, perché non possono più gridare. Ma quanto vi manca gridare a quest'Assemblea «Lamorgese, dimettiti»? Quanto vi manca dispensare facili soluzioni a problemi complessi? Il vostro nervosismo in queste settimane è palpabile e ogni ogni giorno pare che ci sia una gara a chi la spara più grossa. La maggioranza di Governo oggi accusa il MoVimento 5 Stelle di aver mandato in rovina il Paese con il superbonus al 110 per cento, una misura che fino a pochi mesi fa avevate in mente di estendere in ogni ambito, anche ai formicai. Tuttavia, Tuttavia, consentite a voi stessi di usufruire quotidianamente di un superbonus di scemenze a credito illimitato *(Applausi)*, in barba al ruolo istituzionale e di Governo che continuate a svilire. Il Paese continua a soffrire per le vostre mancanze. Siete partiti dal diario di Giorgia, che doveva essere pieno di appunti. quanto pare è rimasto bianco, completamente intatto e candido, perché avete dimenticato di sostituire l'inchiostro della propaganda con quello della concretezza, della coerenza, della serietà e della responsabilità. responsabilità. In altre parole, avete dimenticato di governare. Abbiamo quindi una *Premier* che voleva scrivere un diario delle cose fatte, ma dopo un anno lo riconsegna al Paese in bianco, e abbiamo un Vice *Premier* che, peggio mi sento, si affida a Topolino per consigli su come guidare il Paese; sì, perché così un domani Salvini potrà dare la colpa a Topolino di aver autorizzato lo sforamento del tetto di spesa per il compenso dei dirigenti della società Stretto di Messina, norma che avete inserito vergognosamente in questo testo.

Un altro successo del ministro Salvini. Questo provvedimento è solo un altro mattone, ben inserito nella vostra piramidale e ormai stratificata inadeguatezza. Siete i primi e più efficaci detrattori di voi stessi. Per questo e tanti altri motivi che, signor Presidente, non ho il tempo di illustrare, il MoVimento 5 Stelle voterà

con questo decreto-legge ci accingiamo ad approvare una serie di disposizioni urgenti a tutela degli utenti e in materia di attività economiche e investimenti strategici, permettendo così il raggiungimento di più alti livelli nei servizi offerti e l'avvio di una fase di crescita maggiormente strutturata, in previsione della legge di bilancio ormai imminente. Il provvedimento in esame riguarda materie di particolare rilievo... cerca di rispondere alle esigenze di famiglie e imprese e alle problematiche emerse negli ultimi anni di forte crisi e difficoltà, o quantomeno di mitigarne gli effetti negativi su tutto il Paese. Le novità introdotte da questo decreto riguardano la complessa materia delle licenze dei taxi, nonché gli investimenti strategici nel settore delle infrastrutture, ma anche il caro voli e i prelievi degli extraprofitti delle banche limitati al 2023. Ricordiamo in quest'Aula che le prime cinque banche italiane, nel primo semestre del 2023, hanno già accumulato un margine di interesse di 40 miliardi di euro. di questa tassa andranno all'aiuto per i mutui sulla prima casa e al taglio delle tasse, che diventa fondamentale per la ripartenza economica e per il sostegno alle famiglie e alle imprese di questo Paese, in un momento di così grave difficoltà. Si tratta, come ha ribadito il vice *premier* Matteo Salvini, di una norma di equità sociale. Con l'emendamento del Governo, su indicazione della Lega e del ministro Giorgetti, si salvano le piccole banche, mettendo a riserva questa eventuale partecipazione alla tassa che doveva essere effettuata; ma soprattutto diamo sostegno a chi eroga credito più facilmente alla clientela più piccola e salvaguardiamo i risparmi delle famiglie e delle imprese e non li mettiamo in discussione. Per quanto riguarda il settore dei taxi, viene consentito ai Comuni di rilasciare, in via sperimentale, licenze aggiuntive a carattere temporaneo per l'esercizio del servizio, in favore di chi già sia titolare di licenza, il quale può affidare la licenza aggiuntiva a terzi o gestirla in proprio, anche tramite un sostituto alla guida, nel rispetto di regole ben definite. In materia di caro voli, pensiamo di aver frenato in via definitiva l'asta che si determina in alcune condizioni, quando vi è il massimo delle richieste e un arbitrio che in questo modo non sarà più consentito realizzare. Viene stabilito un tetto massimo per nuove gare dei servizi pubblici per le isole e, per quello che è già vigente, per l'algoritmo che di fatto realizza una sorta di asta dei voli e una prassi commerciale scorretta che porta a pregiudizi per l'utente. Un'altra parte fondamentale del decreto contiene le misure di estensione della *golden power*, importantissima nel caso di trasferimento all'estero di tecnologia particolarmente critica. Anche quando questo trasferimento avvenga infragruppo, si autorizza l'esercizio dei poteri speciali quando atti e operazioni riguardino intelligenza artificiale, macchinari per la produzione di semiconduttori, *cybersecurity*, tecnologia aerospaziale, stoccaggio di energia quantistica e nucleare. Se un'impresa delocalizza nei primi dieci anni di attività, dovrà restituire gli incentivi. Per quanto riguarda l'attrazione degli investimenti esteri, per rafforzare gli strumenti e quanto messo in atto già dall'inizio della legislatura, sarà possibile nominare commissari straordinari per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione, nel caso di investimenti esteri superiori a un miliardo. Si interviene anche sul caro materiali, che sta molto a cuore, soprattutto in questo momento così particolare, per permettere la realizzazione di interventi indifferibili, quali tra l'altro l'alta velocità ferroviaria. Un intervento riguarda anche il settore dell'autotrasporto merci, al fine di andare incontro alla crisi del comparto. Si esclude il settore dalle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), con la conseguente soppressione del contributo annuale da parte degli autotrasportatori. una misura di buona e sana amministrazione, che elimina un onere burocratico a carico della categoria degli autotrasportatori, attribuendo al Ministero delle infrastrutture, con un significativo risparmio di spesa, le funzioni di regolazione del settore.

è un punto importantissimo che vorrei ricordare a quest'Aula, che non è stato citato: il fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni, fortemente voluto dal Ministero delle infrastrutture. E qui ringrazio il vice ministro Rixi per l'attività svolta, soprattutto in Commissione,

50 milioni di euro dal 2023 al 2025. Potranno presentare richieste di contributo i Comuni fino a 5.000 abitanti, per interventi dal costo non superiore a 150.000 euro. La misura interviene anche in modo importante, perché dà sostegno alle piccole comunità e diventa importante rafforzare ed efficientare i piccoli comuni. Abbiamo poi misure sia nel settore vitivinicolo che nel settore riguardante la pesca per quanto riguarda la cattura e lo smaltimento della specie del granchio blu. In tema di efficientamento energetico, viene esteso, dal 30 settembre al 31 dicembre, il termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del superbonus 110 per cento, sulle spese sostenute o su interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti autonome, che, alla data del 30 settembre 2022, avevano già completato i lavori per circa il 30

In questi decenni è cambiato tantissimo il percorso di questa strada, che è sempre più frequentata. L'Anas aveva preparato, dal 1990 in poi, ben cinque progetti, tutti bocciati per i motivi più diversi: ambientali, idrogeologici, consumo del territorio troppo cari. L'ultimo progetto valeva circa cento milioni di euro, ma alla fine non è stato finanziato. Il nuovo progetto della variante è stato presentato a ottobre 2019. Ottenuti i pareri favorevoli di alcuni enti importanti, è mancato il parere del Ministero dei beni culturali, che ha bocciato la proposta per motivi paesaggistici. Nel bando erano presenti in Anas risorse per circa 50 milioni di euro. Con gli aumenti di costi, stimiamo che oggi superino gli 80 milioni di euro. Con l'approvazione, però, dell'emendamento dei relatori, a firma mia e del collega Rosso, presentato all'articolo 19, si mette un punto fermo su questa parte di progettazione da parte del Governo, che dovrà nominare un Commissario straordinario per l'esecuzione della variante di Demonte. Ed è stato messo nero su bianco che la fase realizzativa dell'opera

Abbiamo, inoltre, confermato la grande attenzione per i territori colpiti dalle alluvioni di quest'estate, consentendo alle Regioni, con l'emendamento a prima firma del Presidente del nostro Gruppo, il senatore Romeo, Romeo, di anticipare fino a 235 milioni di euro di interventi per affrontare i danni subiti e a favore delle zone alluvionate. Sono stati inoltre incrementati di 370 milioni per il 2023 i fondi per la ricostruzione. Parliamo di risorse per un totale superiore a mezzo miliardo di euro, immediatamente disponibili per problemi che si sono verificati su più Regioni del nostro territorio nazionale. Si è agito anche per rimuovere gli ostacoli di ordine amministrativo e burocratico, che sono motivo di intralcio allo sviluppo del Paese. Per quanto riguarda l'attività venatoria, vorrei tranquillizzare i colleghi che non è successo nulla di catastrofico. Abbiamo semplicemente fatto fare un passo in avanti al settore, nel recepimento del Regolamento europeo sul divieto di uso delle munizioni di piombo nelle aree umide, con l'obiettivo di dare la certezza del diritto a coloro che praticano attività venatoria. Non dimentichiamo che l'attività di gestione della fauna selvatica contribuisce in modo determinante al contenimento della peste suina africana, una delle piaghe dalle quali il nostro Paese sta cercando di risollevarsi, che non coinvolge solo una Regione, ma coinvolge più territori. Un passo dopo l'altro ci avviciniamo alla legge di bilancio e su ogni provvedimento la maggioranza parlamentare e il Governo hanno dimostrato capacità di dialogo e determinazione molto importanti. Oltre al vice Ministro voglio ringraziare anche i due presidenti delle Commissioni, senatori De Carlo, per il loro impegno nonché i commissari per aver analizzato 550 emendamenti con molta capacità ed attenzione. Termino richiamando comunque l'Aula agli impegni che noi assumiamo nei confronti del Governo e del Parlamento, ringraziando che comunque su ogni provvedimento possiamo intervenire cercando di migliorarlo grazie alla grande disponibilità

Signor Presidente, ascoltando i colleghi della maggioranza si ha l'impressione che forse in questi giorni abbiamo vissuto realtà diverse e analizzato provvedimenti diversi. Siamo all'ennesimo decreto di urgenza, questa volta fatto - devo dire che si vede - ad agosto, sotto l'ombrellone;

è che le principali proposte cosiddette di urgenza sono state emendate dallo stesso Governo in quella che è una vera e propria ritirata. Hanno ragione i colleghi che hanno detto che d'estate si annunciano dei provvedimenti solo per fare qualche *tweet*, per andare sulla stampa, per illudere gli italiani che c'è un tetto al prezzo dei voli o che, in qualche misura, ci saranno 3-4 miliardi da spendere in spese sociali, prese da i cosiddetti extraprofitti delle banche. Dibattiti, prese prese di posizione, rivendicazioni, dopodiché il Governo stesso, per primo, presenta due emendamenti in cui cancella le sue principali proposte. *(Applausi)*. E in più su questo ci mette la fiducia. Secondo me fa bene a farlo perché ci vuole veramente una grande fiducia in un Governo che fa un provvedimento d'urgenza

questo Governo produca un unico grande decreto *omnibus* a puntate, un po' come certe riviste di una volta dove c'erano tante sezioni (la sezione

democratica. Da questo punto di vista il Governo invece insiste nella sua corsa, ma la cosa che ci lascia ancora più perplessi è

è che nei nodi fondamentali, negli stralci fondamentali di intervento delle proposte dell'opposizione, non c'è stato alcuno spazio per una discussione costruttiva. Iniziamo dalle banche; vi era una proposta che ha bruciato in due giorni 10 miliardi alle banche del nostro Paese per produrre eventualmente circa 2 miliardi a metà anno del 2024. Adesso il Governo, in un certo senso una parte di un emendamento (bocciato) del Partito Democratico, propone un incentivo che fa sì che tutti questi extrautili diventino riserve, mentre noi abbiamo proposto che venisse istituito un fondo per dare risposte, come suggerisce la BCE a proposito dei prelievi delle banche, agli utenti, ai clienti, alle famiglie *(Applausi)*, al fondo per la prima casa, alla proposta sulla rateizzazione dei mutui, alla proposta relativa alle prime case per i giovani, alle imprese che hanno visto incrementare i costi dei propri crediti. Nulla di questo è stato approvato, neanche un emendamento, signor Presidente, che proponeva semplicemente di considerare questi possibili impieghi per le entrate eventuali di una tassa che non c'è, che non viene applicata, che è stata annunciata, ma che effettivamente non produrrà nessun gettito spendibile per il sostegno della spesa sociale. Inoltre, vi è un evento abbastanza traumatico nella produzione di questa norma, perché sostanzialmente questa stessa norma, nel momento stesso in cui viene emendata

una riduzione della crescita attesa del PIL, un aumento prospettico della manovra in *deficit* che si vede anche nell'incremento dello *spread*, quindi sostanzialmente un insieme di misure confuse. Voglio citare una norma che ci ha lasciato molto perplessi e che noi riprodurremo nel decreto concorrenza, la cosiddetta norma TIM. Vi è stata chiesta la fiducia per due miliardi e mezzo per operazioni che non sappiamo quali quali saranno. Abbiamo inserito una serie di emendamenti su Telecom Italia perché sappiamo, dal decreto della Presidente del Consiglio dei ministri, che quello è lo sbocco, ma sostanzialmente noi stiamo impegnando miliardi e mezzo di risorse pubbliche per comprare una rete che non sarà una rete complessiva del Paese, non sarà una rete a controllo pubblico, sarà una rete deflazionata *(Applausi)*, vedrà ancora problemi di sicurezza e ridurrà la concorrenza nel Paese e il valore per l'impresa TIM e anche per i suoi azionisti. Una strategia del tutto contraria a quella annunciata nella campagna elettorale dei vostri partiti in cui insistevate sulla sovranità e sulla sicurezza dei dati. state dando il là ad un'operazione che mortifica il valore della rete, che sperpera soldi pubblici senza neanche garantire il controllo. Per quanto riguarda i voli, scusate, voi lo sapete e mi prendete anche in giro, io sono siciliano.

287 del 1990 attribuisce a tale Autorità, anche in questo caso inserendo una innovazione nella legge n. 287 del 1990 che richiederà ancora un intervento perché non si possono modificare i poteri dell'Autorità indipendente solo per un settore, senza coinvolgere, come sosteneva un nostro emendamento, l'Autorità di regolazione del settore. Non possiamo, con tutto il rispetto delle autorità indipendenti, delegare loro la politica industriale. Poi ancora, avete avete fatto un provvedimento in cui sostanzialmente avete stanziato, giustamente, risorse per gli incendi in Sicilia e in Sardegna, ma soltanto fino al 7 agosto, quando sappiamo che gran parte dei danni sono avvenuti dopo. Abbiamo presentato un emendamento per spostare tale data al 30 agosto. Lo chiedo ai colleghi siciliani: come fate a ritornare in Sicilia questo fine settimana e a spiegare a tutti coloro che hanno avuto dei danni nel contesto turistico che questa copertura non c'è stata? La stessa cosa vale per tutti gli emendamenti relativi alla situazione in Emilia Romagna. Continuate a dire che date un sostegno: non è arrivato nulla da quello che ci dicono gli amministratori locali.

industriale. Qui c'è un tema che non riguarda soltanto il Governo e l'azione del Governo nel mettere la fiducia: c'è un problema che riguarda voi, colleghi senatori della maggioranza, che tocca dimostrare l'orgoglio della vostra vita da legislatori. Voi dovete pretendere che il Governo che vi chiede la fiducia abbia fiducia in voi, nelle vostre capacità di istruire un lavoro nelle Commissioni che analizzi le questioni, il merito e i problemi. Oggi questo Governo così lontano dal merito non vi ha chiesto in effetti la fiducia, ma vi sta chiedendo fedeltà e, quando un Governo si muove e si sostiene soltanto sulla fedeltà dei suoi sostenitori, evidentemente non solo non era pronto, ma sta già finendo la sua corsa. Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il decreto-legge n. 104, che oggi è sottoposto alla nostra attenzione, è un provvedimento molto importante, all'interno del quale si affrontano tematiche di grande valenza e di stringente attualità in materia di attività economiche, finanziarie e di investimenti strategici. Ma prevede altresì - come è stato ricordato - alcune disposizioni a tutela degli utenti, quale certamente quella inserita all'interno dell'articolo 1, laddove si affronta un tema molto importante quale quello del caro voli. questa problematica si parla da moltissimi anni, ma al riguardo non c'è stato mai un intervento pragmatico da parte dei Governi che si sono alternati. Lo dico da siciliano che reputa come ritengo anche il collega Nicita - assolutamente offensivo ed eticamente non giustificabile dover pagare un volo Catania-Roma o Palermo-Roma - come sanno meglio di me i colleghi Russo e Sallemi - 1.000 euro, più di quanto si paghi per un Roma-Sidney o un Roma-New York. È opportuno che sappiate che la tratta Catania-Roma, la più trafficata d'Italia, è quella più remunerativa per le compagnie aeree e questo accade perché di fatto in Sicilia non ci sono sono mezzi di trasporto alternativi per poter raggiungere in tempi ragionevoli la Lombardia, il Lazio, il Veneto e le altre Regioni italiane.

al progetto qualificante del Ponte sullo Stretto, fortemente voluto dal Governo Meloni e dal ministro Salvini, dopo cinquantadue anni di parole al vento che sono costate centinaia di milioni di euro, da quando nel 1971 si costituì la società Stretto di Messina. Ebbene, quel percorso di parole al vento finalmente si è concluso e dal 2024 si apriranno i cantieri, nel 2032 si completerà quell'opera di fondamentale importanza non soltanto per la Sicilia e la Calabria, ma per tutta la nostra Nazione.

alcuni Governi hanno tentato di affrontare questa tematica, ma le iniziative, seppur lodevoli dal punto di vista concettuale, non hanno sortito alcun effetto. Penso a quanto è accaduto con il finanziamento di un progetto denominato

perché sono state immaginate procedure farraginose e restrittive. Il Governo Meloni sta affrontando anche questo tema grazie al ministro Salvini, al vice ministro Bignami, in sinergia con la Regione Sicilia, col presidente Schifani e l'assessore Aricò, e queste regole verranno modificate. Tuttavia, nelle more che esse cambino, era importante intervenire su un tema molto sentito all'interno non soltanto della mia Regione e della Sardegna, ma anche di altri contesti territoriali, come quello dell'Emilia Romagna; contesti che hanno vissuto l'eresia del caro voli, laddove, nonostante fossero colpiti da alcune emergenze atmosferiche (mi riferisco all'alluvione di qualche mese fa) con l'interruzione contestuale dei trasporti ferroviari e stradali, hanno registrato anche un prezzo eretico per trasferimenti aerei da parte alcune compagnie aeree nelle tratte da Roma a Bologna. Credo infatti che questo intervento normativo serva anche ad evitare queste assolute eresie. modo reputo opportune ed equilibrate - contrariamente a quanto è stato detto da qualche collega che mi ha preceduto - le misure previste per affrontare un'altra oggettiva criticità, qual è quella delle carenze del sistema di trasporto taxi su gomma.

alla data di pubblicazione del bando. I proventi di questi bandi sono destinati a un fondo che servirà a compensare i titolari di licenza alla data di pubblicazione del bando. Credo che si siano trovate delle soluzioni equilibrate per rispondere a due esigenze fortemente sentite: la prima è quella di tutelare gli utenti all'interno di un

i titolari delle vecchie licenze che in passato hanno investito molte risorse per poterle acquisire. Considero molto importante anche l'intervento previsto all'articolo 4,

laddove sono inseriti incentivi nella forma del credito d'imposta per le imprese che operano all'interno del settore dei semiconduttori

asiatici. Questo è un problema non soltanto politico ed economico, ma è anche geopolitico che viene affrontato con altrettanta determinazione da parte del Governo Meloni. L'articolo 8 prevede l'innalzamento del divieto di delocalizzare per le imprese che hanno ottenuto ingenti finanziamenti per alcuni progetti qualificati, pena la perdita dei finanziamenti ottenuti. E credo che questo sia un intervento normativo che tutela l'interesse nazionale. *(Applausi)*. Stessa cosa è sancita all'interno dell'articolo 13, dove si affronta il tema dei programmi di investimento esteri in territorio nazionale, ma all'interno di settori strategici con investimenti superiori a un miliardo di euro, è prevista la possibilità di nomina di un Commissario straordinario di Governo che possa accelerare le pratiche burocratiche e amministrative, anche attraverso una Conferenza dei servizi. servizi. Importante è anche l'intervento a sostegno dei Comuni in dissesto finanziario, previsto all'articolo 23, con un'anticipazione di liquidità da 100 milioni di euro nel 2024, 2025 e 2026, che faciliti il pagamento dei debiti. Altrettanto importante, infine, è quanto previsto dall'articolo 26 in riferimento all'imposta straordinaria a carico delle banche: una norma che è stata modificata attraverso l'emendamento governativo, mirante a cambiare la base imponibile, ma che ha il grande merito di affrontare un tema molto delicato, quale certamente è quello dei profitti straordinari realizzati dopo l'aumento dei tassi di interesse, fortemente voluto dalla Banca centrale europea. Ricordo a me stesso e a chi ci ascolta che la Banca d'Italia ha sancito qualche mese fa come i tassi di interessi sui mutui abbiano raggiunto il 4,75 per cento. A fronte di questo aumento non c'è stato un contestuale aumento dei tassi applicati nei confronti dei titolari di conti correnti o di conti depositi. Ecco perché era giusto intervenire in tal senso: credo che sia un problema di giustizia sociale che il Governo Meloni ha affrontato in maniera assolutamente qualificante.*(Applausi)*. Siamo quindi in presenza di un decreto-legge che affronta alcune tematiche molto importanti per la nostra Nazione, in maniera pragmatica e altrettanto equilibrata, avendo come stella polare la tutela dell'interesse nazionale che credo rappresenti una discriminante del Governo Meloni, che persegue anche attraverso questo intervento normativo. Questo è il motivo per il quale, con orgoglio, preannunzio il voto favorevole di Fratelli d'Italia su questo importante provvedimento.

la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello. Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

Borgonzoni.

Proclamo il risultato della votazione

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge